di iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia: «Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n 118, recante misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale,

con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'on. Claudio DURIGON dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze. *F.to* Mario Onorevoli colleghi, come è tristemente noto, il 20 agosto scorso è venuto a mancare il senatore Paolo Saviane. Invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio in ricordo del compianto collega, il cui ricordo si farà in maniera più compiuta in una prossima occasione.

Signora Presidente, senatrici e senatori, dopo aver aggiornato il Copasir e le Commissioni esteri e difesa, ritengo fondamentale continuare insieme al ministro Guerini in quest'Aula un intenso e proficuo dialogo con il Parlamento. Prima ancora che come parlamentari o membri del Governo, quanto sta accadendo in Afghanistan ci chiama in causa come donne e uomini. Le immagini strazianti dei profughi e le aspettative di pace e sviluppo di un intero popolo ribaltate in pochi giorni non ci lasciano indifferenti. Non ci lascia certo indifferenti la prospettiva che i progressi faticosamente raggiunti in vent'anni, soprattutto per le donne, possano essere cancellati. Lavoriamo perché ciò non avvenga rimanendo al fianco del popolo afgano. Questa crisi ripropone l'esigenza di un multilateralismo più efficace ed inclusivo e al tempo stesso la necessità di una forte coesione europea e di un'autonomia strategica e operativa dell'Unione nell'alveo delle nostre consolidate alleanze in piena sinergia con i *partner*. La risposta agli eventi delle ultime settimane in Afghanistan ha richiesto sin da subito uno sforzo di coordinamento internazionale senza precedenti. Sicurezza, gestione dei flussi migratori, contrasto al terrorismo e narcotraffico, assistenza umanitaria e tutela dei diritti universali, sono sfide che possono essere affrontate solo con un approccio a più dimensioni. Da settimane siamo in costante contatto con i principali interlocutori internazionali utilizzando tutti i formati disponibili, dall'Unione europea al G7, dalla NATO alle Nazioni Unite. È prevista domani una nuova riunione a livello ministeriale con un formato ampiamente inclusivo copresieduta dal segretario di Stato Blinken. Anche a livello bilaterale i contatti sono continui, del presidente Draghi e i miei. Oltre che con i colleghi europei, ho avuto nelle ultime settimane colloqui telefonici e incontri anche con i miei omologhi di Stati Uniti, Russia, Cina, Canada e India. Poche ore fa sono rientrato da una missione nella regione, che mi ha portato in Uzbekistan, Tagikistan, Qatar e Pakistan. Con i vari interlocutori ho discusso della stabilità regionale, contrasto al terrorismo e lotta al traffico di droga. Abbiamo deciso di sviluppare una collaborazione bilaterale su due fronti: maggiore sinergia tra le nostre *intelligence* e assistenza umanitaria ai rifugiati, con l'obiettivo di costruire un percorso comune per proteggere la popolazione civile e i soggetti più vulnerabili. Nei prossimi giorni avvieremo i necessari contatti operativi. Crediamo nella necessità di coinvolgere tutti gli attori internazionali che possano contribuire alla definizione di una strategia sostenibile nei confronti dell'Afghanistan. Come Presidenza di turno abbiamo proposto la piattaforma del G20, più ampia e inclusiva, per affrontare le principali sfide del *dossier* afghano. Stiamo verificando condizioni, modalità e tempistiche per un vertice straordinario dedicato all'Afghanistan che potrebbe essere preceduto da riunioni preparatorie dei Ministri degli esteri. L'importanza di un coinvolgimento del G20 è stata riconosciuta anche nella riunione informale dei Ministri degli esteri dell'Unione europea cui ho partecipato la settimana scorsa in Slovenia. Una settimana fa si è chiusa la prima fase, quella emergenziale, in risposta ad un succedersi degli eventi ben più rapido di quanto l'intera comunità internazionale avesse previsto. La priorità è stata l'evacuazione: nel giro di pochi giorni abbiamo messo in salvo e trasferito in Italia 5.011 persone, di cui 4.890 afghani, più della metà donne e bambini, tra quanti hanno collaborato con le istituzioni italiane e appartengono a categorie vulnerabili. Il ponte aereo ininterrotto, realizzato grazie alla sinergia fra tutti gli alleati, ha consentito di far uscire dall'Afghanistan complessivamente oltre 120.000 persone, compresi interi nuclei familiari. L'Italia, tra i Paesi europei, ha evacuato il maggior numero di cittadini afghani. Il ministro Guerini potrà fornire maggiori dettagli, lasciatemi però ribadire la profonda gratitudine di noi tutti alle Forze armate, al corpo diplomatico e all'*intelligence.* Il successo di un'operazione condotta contro il tempo e in condizioni estreme è frutto di uno stretto coordinamento tra i comparti esteri, difesa e *intelligence*, dell'impegno instancabile e coraggioso dei nostri diplomatici, militari, della collaborazione con le organizzazioni della società civile, ma anche del sostegno dei nostri *partner* regionali internazionali, in primo luogo Stati Uniti, Qatar, Kuwait, Pakistan, che non hanno esitato ad attivare procedure straordinarie per aiutarci. A questi Paesi e a questi Governi esprimiamo sincera riconoscenza. Conclusa l'emergenza, abbiamo ora avviato una fase nuova di pianificazione e gestione della crisi. L'Italia continuerà ad aiutare gli afghani che intendano lasciare il Paese e ne abbiano titolo. Le operazioni dovranno naturalmente essere condotte in modo diverso, data la partenza definitiva dei contingenti militari e la chiusura allo stato attuale della nostra ambasciata a Kabul. Ci stiamo muovendo su più fronti: da un lato lavoriamo con i Paesi che collaboreranno per la futura gestione dell'aeroporto di Kabul, in particolare Qatar e Turchia; il Ministro degli esteri qatarino mi ha aggiornato sulla assistenza tecnica fornita per il ripristino dell'operatività dello scalo; già da qualche giorno sono stati riavviati i voli interni. Il Ministro si è anche mostrato fiducioso sul ripristino delle condizioni di sicurezza dell'aeroporto. Dall'altro lato, stiamo interagendo con i Paesi limitrofi per l'individuazione di percorsi umanitari che consentano l'espatrio per quanti arrivano dall'Afghanistan via terra. Oltre al tema delle evacuazioni, il confronto multilaterale prosegue su base quotidiana con riunioni a livello politico e tecnico su altri fondamentali profili, in primo luogo sulla presenza diplomatica a Kabul dopo la chiusura temporanea della maggior parte delle ambasciate. Ora abbiamo deciso di trasferire la nostra ambasciata a Doha come ufficio diplomatico, in linea con quanto facendo altri Paesi come Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Canada e in prospettiva Olanda e Spagna. di parlare con il mio omologo qatarino, che ha confermato massima collaborazione. Ci sembra un'opzione efficace perché consente contatti con potenziali interlocutori, con i Paesi dell'area e con i nostri *partner* che hanno già dislocato in Qatar i propri punti di rappresentanza competenti per l'Afghanistan. Stiamo anche riflettendo sulla creazione di una presenza congiunta in Afghanistan, un nucleo formato da funzionari di più Paesi sotto l'ombrello dell'Unione europea o eventualmente delle Nazioni Unite, con funzioni prevalentemente consolari e che serva da punto di contatto immediato. Si tratterebbe di una soluzione innovativa, per la quale sarà necessario un efficace coordinamento preventivo sia per gli aspetti di sicurezza, sia per la necessità di definire un mandato chiaro. Qualunque modalità prescelta dovrà in ogni caso essere inclusiva, condivisa con tutti i Paesi potenzialmente interessati a contribuire. Il secondo tema al centro del coordinamento internazionale riguarda l'atteggiamento da mantenere nei confronti dei talebani e più in generale della futura dirigenza afghana. L'approccio dell'Italia si inserisce anzitutto nel solco di un'impostazione condivisa a livello europeo, ne abbiamo discusso la scorsa settimana nella riunione informale dei Ministri degli esteri dell'Unione in Slovenia. Per poter proseguire nel nostro sostegno al popolo afghano, abbiamo convenuto che i talebani vanno giudicati sulla base delle loro azioni e non delle dichiarazioni, azioni che intendiamo misurare in base a cinque parametri. il ripudio del terrorismo e la cooperazione del contrasto al narcotraffico. Due: il rispetto dei diritti umani (in particolare di donne e minoranze), dello Stato di diritto e della libertà dei *media*. l'istituzione di un Governo inclusivo e rappresentativo. Quattro: la garanzia di incondizionato e sicuro accesso umanitario per le organizzazioni internazionali, in particolare delle Nazioni Unite. il rispetto dell'impegno assunto, volto ad assicurare il libero passaggio a coloro che intendano lasciare il Paese, in linea con la risoluzione n. 2593, approvata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite lo scorso 30 agosto. di concetti che trovano ampia condivisione anche nei Paesi che ho visitato in questi giorni. Certo, ciò che stiamo vedendo in Afghanistan in queste ore non è affatto incoraggiante. Sulla base di queste condizioni fondamentali, il nostro approccio deve unire al pragmatismo sul piano operativo la fermezza sui principi. Vigilare sul rispetto di queste condizioni e calibrare, di conseguenza, il nostro comune atteggiamento nei confronti delle autorità afghane ci consentirà anche di utilizzare efficacemente le leve di cui disponiamo nei loro confronti. Una delle leve più importanti a disposizione è l'assistenza economico-finanziaria. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che l'Unione europea è il primo erogatore di aiuti allo sviluppo e, per questo, un'azione concertata anzitutto a livello europeo è particolarmente cruciale. Il terzo punto su cui è imprescindibile un'azione coordinata è quello della stabilità regionale e della sicurezza internazionale. Il Ministro degli esteri tagiko, ad esempio, mi ha trasmesso la preoccupazione e il grave senso di vulnerabilità del suo Paese lungo il confine con l'Afghanistan. Per sorvegliare questa frontiera il Tagikistan ha richiamato in servizio attivo nell'esercito oltre 20.000 riservisti. Dobbiamo prevenire il rischio che la crisi afghana abbia un impatto negativo destabilizzante sui Paesi limitrofi, con implicazioni che potrebbero andare ben oltre la dimensione regionale. Mi riferisco anzitutto al contrasto al terrorismo. Gli attacchi del 26 agosto scorso all'aeroporto internazionale di Kabul, con il loro pesante bilancio di vittime e feriti, testimoniano come il terrorismo rappresenti una minaccia concreta e immediata. Oltre all'Isis-Khorasan, che ha rivendicato gli attacchi, nel Paese operano gruppi estremisti affiliati ad al-Qaeda con cui i talebani mantengono talvolta un approccio ambiguo. Abbiamo contrastato il terrorismo in Afghanistan per vent'anni e siamo riusciti a raggiungere importanti risultati anche al costo della vita di 54 militari italiani, cui vanno il nostro ricordo e la nostra gratitudine.

Il Paese non può e non deve tornare a essere un rifugio sicuro per i terroristi. Dobbiamo stringere alleanze e coinvolgere tutti gli attori (specie quelli della regione) che condividono questa stessa preoccupazione, oltre a Russia e Cina. Altrettanto importante sotto il profilo della sicurezza è la lotta al traffico di stupefacenti. Il narcotraffico è un'importante fonte di finanziamento dei talebani. La produzione afghana di oppio da cui si ricava l'eroina rappresenta circa l'85 per cento di quella mondiale. Stiamo valutando iniziative nel settore della lotta al narcotraffico in raccordo con le competenti agenzie delle Nazioni Unite, a partire dall'Ufficio per il controllo della droga e la prevenzione del crimine. L'Italia intende contribuire alla gestione internazionale della crisi afghana con proposte concrete, articolate in un piano di azione nazionale a sostegno del popolo afghano. Si tratta di uno sforzo corale di tutte le nostre amministrazioni che dovrà coinvolgere anche la società civile e gli enti territoriali, il cui contributo è indispensabile. La sua realizzazione si gioverà anche di risorse e strumenti internazionali, ad esempio dell'Unione europea e delle Nazioni Unite. Il piano che ho già condiviso nelle sue linee fondamentali in Consiglio dei ministri è per sua natura in evoluzione e dovrà essere progressivamente adattato agli sviluppi sul terreno e alle esigenze che dovessero manifestarsi. La prima riunione tra amministrazioni per la definizione del piano, coordinata dalla Farnesina, si è tenuta una settimana fa e ha consentito di individuare i cinque pilastri su cui poggia questa strategia nazionale. Il primo riguarda l'assistenza umanitaria. Il segretario generale Guterres ha convocato per lunedì prossimo una conferenza internazionale per discutere dell'emergenza Afghanistan. L'attuale crisi si è aggiunta alle conseguenze di un conflitto protratto, agli effetti della siccità e della carestia e all'impatto della pandemia. Un afghano su tre ha problemi per mangiare, una situazione che riguarda metà dei bambini al di sotto dei cinque anni, mentre gli sfollati interni sono oltre 550.000 dall'inizio dell'anno. Dobbiamo fare ogni sforzo per evitare una catastrofe umanitaria. Giovedì scorso, su mia proposta, il Consiglio dei ministri ha destinato 120 milioni di euro a iniziative di resilienza a favore della popolazione afghana, all'assistenza ai rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché alla partecipazione italiana all'attuazione di programmi internazionali di risposta alla crisi in Afghanistan. Si tratta di fondi che erano originariamente destinati alla formazione delle forze di sicurezza afghane nell'ambito della delibera missioni. Auspico di nuovo il sostegno del Parlamento per autorizzare quanto prima l'attribuzione di queste risorse da utilizzare entro fine anno. Stiamo rivedendo la programmazione della cooperazione allo sviluppo per riorientare i fondi previsti per l'Afghanistan anche in questo caso verso interventi a carattere umanitario. Le risorse per il 2021 verranno portate da 21 a 31 milioni di euro complessivi, destinandole a iniziative per l'assistenza alimentare, per servizi di salute materno-infantile e per la lotta alla malnutrizione infantile e, in generale, per la tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione come donne, minori e sfollati interni. Gli interventi potranno aver luogo sul canale multilaterale, tenendo conto dell'effettiva possibilità per le organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite o della famiglia della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa di operare in sicurezza in Afghanistan e nei Paesi limitrofi. Ci stiamo adoperando perché alle organizzazioni internazionali sia assicurato l'accesso umanitario pieno, sicuro e senza ostacoli al Paese, garantendo che gli aiuti arrivino ai diretti ed effettivi destinatari. Ne ho discusso, nei miei contatti, con il Segretario generale delle Nazioni Unite e con l'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati Filippo Grandi. La presenza e operatività in Afghanistan delle agenzie specializzate ONU è la nostra priorità. Continuiamo a lavorare anche nell'ambito del programma COVAX, perché prosegua con sempre maggiore efficacia l'azione di risposta alla pandemia in Afghanistan, dove sono state già consegnate 2,5 milioni di dosi. Tra le categorie più bisognose di assistenza umanitaria vi sono sfollati e rifugiati. Il secondo pilastro del piano nazionale è, dunque, la messa a punto di una risposta strutturale al flusso di rifugiati dall'Afghanistan verso i Paesi vicini e potenzialmente verso l'Europa. Per gli afghani in condizione di particolare vulnerabilità, soprattutto donne e minori, stiamo lavorando per verificare la possibilità di attivare percorsi sicuri in direzione dei Paesi limitrofi, anche con l'ausilio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni. In Tagikistan ho incontrato i rappresentanti di UNHCR per constatare direttamente la situazione sul terreno. In Qatar ho visitato una delle strutture di prima accoglienza e transito di civili dall'Afghanistan, toccando con mano l'importante sforzo messo in campo dal Paese in coordinamento con gli Stati Uniti per facilitare le operazioni umanitarie. In Pakistan, dove abbiamo istituito in ambasciata una *situation room* per la gestione dei profughi afghani, ho tenuto a visitare la frontiera con l'Afghanistan a Torkham. Dai sopralluoghi che ho svolto e come mi hanno confermato gli interlocutori della cooperazione allo sviluppo sul campo, almeno per il momento, dal punto di vista dei flussi migratori la situazione rimane sotto controllo, ma il rischio è che la crisi economica e alimentare, anche in vista dell'inverno, possa innescare flussi più ampi. Tutti i rappresentanti dei Governi che ho incontrato mi hanno manifestato maggior preoccupazione per il rischio di proliferazione della minaccia terroristica. Nei giorni scorsi si sono verificati alcuni attentati al confine tra Afghanistan e Pakistan. Proprio per questo abbiamo deciso di rafforzare il coordinamento tra le nostre *intelligence*. Ho istituito un tavolo di coordinamento con le organizzazioni della società civile sull'accoglienza in Italia e sull'assistenza umanitaria ai rifugiati afghani nei Paesi dell'area. Il tavolo, che tornerà a riunirsi il 9 settembre, presieduto dalla vice ministra Marina Sereni, potrà fornire un importante valore aggiunto per la messa a sistema di proposte e capacità. Mobiliteremo il fondo della Farnesina per le migrazioni al fine di sviluppare attività mirate a rafforzare le capacità dei Paesi vicini di gestione dei flussi migratori e accoglienza di migranti e rifugiati. Le priorità sono l'assistenza alle donne, la formazione in materia di diritti umani, la lotta ai trafficanti di esseri umani. L'obiettivo è quello di sostenere istituzioni e comunità locali, ma va inserito nell'ambito di una più ampia strategia di gestione dei flussi migratori che l'Europa è chiamata a mettere in campo. Intendiamo infatti utilizzare il più possibile strumenti di portata europea. Chiederemo l'inserimento dell'Afghanistan come Paese prioritario nel programma di reinsediamento dei rifugiati finanziato tramite il Fondo per l'asilo, la migrazione e l'integrazione dell'Unione europea. Su mia iniziativa, l'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati Grandi è stato invitato al Consiglio esteri informale dell'Unione europea, riunitosi, come ricordavo, la settimana scorsa per riflettere su una strategia d'azione complessiva per fronteggiare la crisi afghana nei suoi diversi aspetti politici, securitari, umanitari e migratori. Leggere la crisi afghana solo attraverso la lente del rischio migratorio è riduttivo e sarebbe un errore anzitutto politico; tuttavia, alla luce delle conseguenze che la situazione umanitaria potrebbe avere a breve e medio termine, è necessario garantire la massima condivisione europea dell'impatto migratorio. A fronte delle esitazioni di alcuni Stati membri, riteniamo necessaria una visione più ambiziosa e coraggiosa del ruolo che l'Unione può giocare, anche assumendo su di sé costi più elevati. Il terzo pilastro del piano d'azione italiano include le iniziative formative. Mi riferisco, ad esempio, alle borse di studio o all'accoglienza presso le università italiane di studentesse e studenti afghani. Il Ministero dell'università e della ricerca ha già avviato una ricognizione capillare presso tutti gli atenei a tal riguardo. Stiamo inoltre lavorando per estendere agli studenti afgani il progetto University corridors for refugees (Unicore), che prevede la creazione di corridoi universitari di studio e integrazione per studenti rifugiati. La Farnesina assicurerà massima collaborazione nella predisposizione di questi percorsi, valorizzando il diritto allo studio come strumento di accoglienza e integrazione e mettendo a frutto quanto sperimentato con successo negli ultimi anni. Numerose sono le manifestazioni di solidarietà della società civile italiana nei confronti delle studentesse e degli studenti afghani. La Farnesina, in raccordo con le altre amministrazioni, ha intrapreso un'azione di razionalizzazione e coordinamento dei diversi tipi di offerte da università, fondazioni e organizzazioni non governative e privati, per canalizzarle verso progetti concreti per l'accoglienza in Italia di studenti afghani. A livello scolastico, il Ministero dell'istruzione ha già messo allo studio le modalità più opportune per assicurare l'erogazione di servizi formativi a favore dei minori afghani giunti in Italia, molti dei quali non conoscono la nostra lingua. Il quarto pilastro riguarda le iniziative per i diritti umani, con particolare attenzione alle donne. Intendiamo promuovere nei *fora* internazionali, a cominciare dalle Nazioni Unite, iniziative appropriate a tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali degli afghani. Lavoreremo per cercare di costruire un consenso in ambito Consiglio per i diritti umani per l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio anche attraverso la promozione di una dichiarazione congiunta nel corso dell'imminente quarantottesima sessione del Consiglio, che comincerà lunedì prossimo. Stiamo anche lavorando all'organizzazione di un evento sulla condizione e sui diritti delle donne in Afghanistan in occasione della prossima settimana ministeriale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Vogliamo inoltre mobilitare le risorse assegnate al quarto Piano d'azione nazionale per l'attuazione dell'agenda donne, pace e sicurezza delle Nazioni Unite, includendovi iniziative per l'Afghanistan. Il quinto pilastro è relativo alle iniziative politico-diplomatiche. È l'elemento centrale perché consente la progressiva messa a punto di una strategia condivisa con i *partner* internazionali e crea i presupposti per facilitarne la realizzazione. Ho già riferito sull'azione che come Italia stiamo portando avanti, a cominciare dal presidente Draghi, nei diversi *fora* internazionali e nei contatti bilaterali. Più in generale, in prospettiva, l'esperienza afghana deve farci riflettere soprattutto in quanto Paesi membri dell'Unione e della NATO. Appare oggi ancor più evidente la necessità di potenziare e mettere a frutto gli strumenti della politica di sicurezza e difesa comune dell'Unione europea. «L'Unione europea ha dimostrato, di fronte alla pandemia e alle sue conseguenze sul piano economico e sociale, una capacità di reazione efficace e tempestiva. Le azioni intraprese, sia sul terreno delle campagne di vaccinazione sia sul terreno del sostegno alle crisi sociali e alla ripresa economica, confermano la bontà delle scelte effettuate in direzione di una sovranità condivisa a livello continentale Analogo impegno deve riguardare ora il contributo dell'Unione europea alla causa della pace dello sviluppo, della sicurezza e della stabilità internazionale». Sono le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono convinto che come europei dobbiamo poter disporre di capacità operative per fronteggiare le situazioni critiche che minacciano i nostri interessi e la nostra stabilità. A quest'obiettivo stiamo lavorando attraverso la messa a punto di una bussola strategica. Voglio dirlo con chiarezza: crediamo nella necessità dell'autonomia strategica europea, ma anche nella complementarità tra politica di sicurezza e difesa comune e Alleanza atlantica. Tra i due aspetti c'è non contraddizione, ma sinergia. Anche in ambito NATO abbiamo deciso di condurre un'analisi onesta e approfondita sulle lezioni apprese con la conclusione della missione Resolute support. Avevamo già lanciato una riflessione di ampio raggio sul futuro della NATO, chiamata NATO 2030, che include anche una revisione del cosiddetto concetto strategico: una riflessione e una revisione rese ancor più necessarie e urgenti dopo i tragici fatti in Afghanistan e a cui l'Italia deve contribuire in maniera sostanziale. Presidente, senatrici e senatori, tutti gli sforzi nazionali e internazionali convergono in questo momento su un obiettivo comune e prioritario: preservare i progressi in termini di diritti umani e libertà civili che la società afghana ha compiuto nell'ultimo ventennio, un patrimonio di valori e capitale umano costruito con grandi sacrifici e investimenti. Non possiamo permettere che vada disperso. Abbiamo sostenuto lo sviluppo della rete infrastrutturale con la costruzione di strade che collegano Kabul all'interno del Paese. Abbiamo riabilitato ospedali e costruito pozzi e sistemi idrici. Nel 2005 appena il 23 per cento della popolazione aveva accesso all'elettricità, nel 2017 il 98 per cento. Le infrastrutture sono cruciali per lo sviluppo, ma quanto si è andato formando nelle menti e nei cuori degli afghani lo è ancor di più ed è più difficile da smantellare. La società afghana oggi ha raggiunto un livello di connessione che rende impensabile tornare a una situazione di chiusura e isolamento analoga a quella di un ventennio fa. Attraverso l'UNESCO abbiamo ripristinato la Educational radio and television (ERTV), che ha fornito al Ministero dell'educazione uno strumento per condurre programmi di formazione ed educazione a distanza. Grazie al nostro impegno e a quello di nostri *partner* e alleati, il tasso di alfabetizzazione dei giovani nel 2018 ha raggiunto il 65 per cento, secondo i dati Unicef. La stessa organizzazione internazionale ci dice che in vent'anni il numero dei bambini a scuola è passato da 1 milione La mortalità sotto i cinque anni si è più che dimezzata: da 128 bambini ogni 1.000 del 2000 a 60 nel 2019; così come si è più che dimezzato il tasso di mortalità materna, passando dalle 1.450 donne decedute nel 2000, ogni 100.000 bambini nati vivi, alle 638 del 2017. Tra il 2001 e il 2018 il tasso di iscrizione femminile nella scuola primaria è balzato da un valore prossimo allo zero a oltre l'80 Le donne sono diventate una parte importante della forza lavoro afghana, arrivando ad occupare oltre un quarto dei seggi in Parlamento. Anche l'aiuto dato ad alcune calciatrici di Herat per farle arrivare in Italia, per cui ringrazio gli enti e le organizzazioni che hanno collaborato, ci ricorda gli spazi che le donne afghane hanno saputo conquistare in questi anni. La libertà di fare sport è tra i semi che abbiamo piantato e che dobbiamo continuare a coltivare. In vent'anni abbiamo contribuito a formare una generazione con una diversa visione della società, basata sui diritti fondamentali di ciascun individuo. Sono quella visione e quella forza che spingono ora donne coraggiose a manifestare a Herat come a Kabul. Non abbandonare il popolo afghano è un nostro interesse e soprattutto un nostro dovere morale. *(Applausi)*.

Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, mi permetterete di rivolgere fin da subito un pensiero riconoscente alle nostre Forze armate per lo straordinario impegno, la grande professionalità e la profonda umanità che ancora una volta hanno dimostrato nell'affrontare la crisi afghana. *(Applausi)*. Sono certo di interpretare in questo doveroso omaggio anche il vostro sentimento. Nell'accogliere a Ciampino il rientro dell'ultimo volo, insieme ai Sottosegretari e ai Presidenti delle Commissioni difesa, ho detto loro che gli italiani sono orgogliosi della straordinaria impresa umanitaria che hanno condotto e che ha reso onore al nostro Paese. Dopo il collega di Maio, che voglio qui ringraziare per l'intensa collaborazione di queste settimane, articolerò il mio intervento sugli sviluppi della crisi afghana con l'obiettivo di illustrare le azioni messe in campo dalla Difesa e di condividere una chiave di lettura per quanto avvenuto e una chiave interpretativa rispetto ai possibili sviluppi della situazione e delle sue ripercussioni sul futuro della politica di difesa e sicurezza nel contesto dello scenario geopolitico attuale. Nel ripercorrere brevemente le azioni attuate dalla Difesa all'indomani dell'annuncio della conclusione della missione della NATO, vi riporto oggi il consuntivo finale dell'operazione di evacuazione dei cittadini afghani, rimandando per i dettagli alle mie comunicazioni dello scorso 24 agosto alle Commissioni congiunte esteri e difesa. L'operazione Aquila omnia ha portato in Italia 5.011 persone, comprensive del personale della nostra ambasciata, e altri cittadini italiani, di cui 4.890 afghani. Siamo di fronte a un numero decisamente superiore a quello dei collaboratori diretti dei nostri contingenti, della nostra missione diplomatica e dei loro familiari, dal momento che le attività di trasporto hanno riguardato anche attivisti dei diritti umani e dei diritti delle donne, giornalisti, membri delle istituzioni e collaboratori delle organizzazioni non governative italiane presenti sul territorio in questi anni, individuati con criteri analoghi e condivisi con gli altri Paesi alleati. un'operazione prettamente militare, che ha comportato un notevole sforzo organizzativo ed operativo, sotto la guida del comando operativo di vertice interforze, in uno scenario difficile e a tratti non permissivo; un'operazione complessa: sono stati eseguiti novanta voli attraverso un consistente spiegamento di mezzi aerei, tra velivoli C-130 e aerei KC-767. La presenza a Kabul di una *joint evacuation task force*, composta da 119 militari, ha assicurato la cornice di sicurezza, il supporto sanitario e le funzioni di comando, controllo e comunicazioni strategiche, in stretto ed efficace coordinamento con il personale diplomatico e militare della nostra ambasciata. La Difesa, all'interno di una cornice organizzativa distribuita in Italia e in teatro operativo, ha visto impegnato un dispositivo di oltre 1.500 unità per attività di trasporto, logistiche e di supporto all'accoglienza e gestione dei rifugiati (per quest'ultima esigenza sono state messe a disposizione anche strutture militari). Permettetemi di dire che si è trattato di un'impresa straordinaria, merito innanzitutto delle donne e degli uomini in divisa, che hanno operato con dedizione e professionalità. Certamente non è il caso di fare classifiche - non mi appassionano neanche - ma credo sia giusto registrare che l'Italia è risultata il Paese dell'Unione europea che ha evacuato il maggior numero di cittadini afghani, grazie al lavoro congiunto delle diverse articolazioni dello Stato coinvolte. Tutte queste attività sono state svolte, inoltre, in stretto coordinamento con gli alleati attraverso un'efficace e reciproco supporto. Voglio evidenziare principalmente la collaborazione con Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Germania, insieme ai quali siamo stati in grado di far fronte anche alle ulteriori richieste di trasporto presentate dall'Unione europea e da altri Paesi. A loro intendo rivolgere, anche in questa sede, il mio più sincero ringraziamento. Come ha già sottolineato il collega Di Maio, altrettanto fondamentali sono stati i contributi dei nostri *partner* regionali, come Qatar, Kuwait e anche Pakistan; questa disponibilità è il frutto di solidi rapporti bilaterali particolarmente significativi anche sul piano tecnico-militare. Su richiesta di Washington, abbiamo reso disponibili le basi di Aviano e Sigonella per il transito dei civili afghani verso gli Stati Uniti. Infine, nell'ambito dell'Alleanza atlantica abbiamo offerto assetti di polizia militare, sanità e *team* specializzati nella cooperazione civile e militare e nel controllo dello spazio aereo, per contribuire all'attività che la NATO potrà decidere di condurre sul proprio territorio per supportare ulteriori attività di accoglienza e supporto umanitario. Le immagini drammatiche dell'aeroporto di Kabul sono ancora davanti ai nostri occhi. Alla soddisfazione dell'impresa portata a termine si affiancano il forte rammarico e la preoccupazione per le persone che non sono riuscite a partire e che aspirano a costruirsi un futuro fuori dall'Afghanistan; anche per questo, la Difesa assicurerà la piena disponibilità per la condotta di eventuali ulteriori attività di evacuazione, secondo modalità e tempistiche che necessariamente dovranno essere ponderate e coordinate nel quadro delle iniziative politico-diplomatiche illustrate poco fa dal ministro Di Maio. L'evoluzione della situazione in Afghanistan ha colto di sorpresa l'intera comunità internazionale, per la rapidità con cui è mutato il contesto politico e militare e per i conseguenti e drammatici risvolti umanitari. Esisteva la consapevolezza comune del rischio di una offensiva talebana nella fase immediatamente successiva al ritiro. Ma, allo stesso tempo, la NATO e la maggior parte degli analisti stimavano che l'efficacia delle forze di sicurezza afghane sarebbe stata perlomeno sufficiente a contenerla: una stima basata sulla larga superiorità numerica delle forze afghane, sulla disponibilità adeguata di equipaggiamenti e sulle valutazioni positive in merito all'operato e alla preparazione dei militari locali, che negli anni più recenti avevano dimostrato una capacità operativa autonoma, frutto soprattutto dell'impegno nelle attività di addestramento svolte dalle forze NATO anche in situazioni complesse. È tuttavia evidente come le cose non siano andate secondo le attese. I talebani si sono mossi per acquisire rapidamente obiettivi di elevata valenza operativa e tattica, come i varchi di confine, i principali centri abitati e le vie di comunicazione verso la capitale: un risultato decisamente agevolato dalla quasi inesistente resistenza delle forze di sicurezza e difesa afghane che, in alcuni casi, non hanno impegnato in combattimento gli avversari, con una condotta non prevedibile e inaspettata per le sue modalità e per le forze in campo. Ci si deve chiedere, dunque, che cosa sia successo e cosa non abbia funzionato. Stiamo parlando di forze armate ben addestrate e ben equipaggiate che, nel corso degli anni, si sono distinte combattendo coraggiosamente, con grandi sacrifici e numerose perdite, contro i talebani, Al Qaeda e Isis. Se gli accordi di Doha e la conclusione della missione Resolution support possono avere avuto un impatto da un punto di vista motivazionale, le ragioni dello sfaldamento delle forze di sicurezza sono da ricercare innanzitutto nella diretta conseguenza di una evidente mancanza di coesione e in uno scarso senso d'identità, ascrivibile soprattutto all'atteggiamento della *leadership* repubblicana che, per diversi motivi, non è stata in grado di svolgere quel ruolo di guida autorevole e rappresentativa che la situazione richiedeva. Questa è una delle prime e più importanti lezioni che, secondo me, dobbiamo assumere ed approfondire dopo l'esperienza condotta in Afghanistan. La decisione della conclusione della missione Resolution support è stata condivisa in ambito NATO, naturalmente all'interno di un confronto che ha visto accenti diversi tra gli alleati, ma anche la volontà di essere coerenti con il valore della coesione dell'Alleanza. Ho già avuto modo di ricordare che, durante la ministeriale nato dello scorso febbraio, avevo rappresentato la necessità di valutare la conferma della presenza delle forze dell'Alleanza anche oltre alla scadenza del 1° maggio, prevista dagli accordi stipulati dall'amministrazione americana. Già allora, il raggiungimento delle condizioni politiche di sicurezza previste dall'accordo appariva lontano dall'essere soddisfatto, visti lo stallo dei colloqui, l'aumento significativo degli attacchi alle forze di sicurezza afghane e gli assassinî mirati di rappresentanti delle istituzioni, dei *media* e della società civile. Abbiamo sempre ritenuto che il dialogo intra afghano e il mantenimento delle istituzioni repubblicane fossero le condizioni indispensabili per il futuro del Paese, ribadendo il nostro orientamento, condiviso anche da altri Paesi europei, circa l'esigenza di correlare le decisioni sulla conclusione definitiva della missione a progressi tangibili di queste condizioni. La difficoltà a raggiungerle ha fatto prevalere, nelle valutazioni dell'amministrazione americana, la scelta di associare il rientro a un approccio temporale, *timebased*, fissando la conclusione della missione Resolution support al 1° maggio e articolando il rientro delle forze entro la data fortemente simbolica dell'11 settembre. Chiaramente, questo cambio di impostazione, a causa del venir meno delle capacità operative, critiche e funzionali al mantenimento del quadro di sicurezza generale dell'intera missione di addestramento e supporto, ha determinato condizioni tali per cui nessun altro Paese alleato poteva rimanere in Afghanistan. Si è arrivati, di conseguenza, al *meeting* straordinario dello scorso 15 aprile, nel quale - come ho detto - pur nella diversità degli accenti tra gli alleati, abbiamo assunto assieme questa decisione, appunto in coerenza con il valore fondante, irrinunciabile e da preservare della coesione dell'Alleanza. Signor Presidente, senatrici e senatori, la cronaca degli ultimi giorni non può e non deve far dimenticare l'impegno nazionale di questi vent'anni nella più grande operazione militare dal termine della Seconda guerra mondiale. Naturalmente, siamo ben consapevoli che i fatti accaduti hanno reso palesi alcuni significativi punti critici, su cui tornerò, ma non possiamo avviare alcuna riflessione su quanto avvenuto senza ricordare le ragioni della missione e anche i risultati conseguiti. All'indomani del tragico attacco alle Torri gemelle nel 2001, a seguito dell'invocazione dell'articolo 5 del Trattato Nord Atlantico, siamo intervenuti con i nostri alleati per combattere il terrorismo globale, che aveva trovato, proprio in Afghanistan, un rifugio sicuro. Aver scelto di agire, di dare il nostro contributo concreto nella lotta contro una minaccia imminente, diretta a tutto l'Occidente e ai suoi valori, è stata una scelta non solo doverosa ma soprattutto giusta. La presenza di Al Qaeda nel Paese è stata resa inefficace; di questo dobbiamo riconoscere il merito, senza alcun dubbio, alla NATO, ai nostri 50.000 militari che si sono avvicendati in questi vent'anni. Prima di tutto per loro dobbiamo ricordare sempre le ragioni della nostra partecipazione, in particolare per i nostri 54 caduti e per gli oltre 700 feriti, cui va il nostro grato e deferente pensiero. Ricorderemo sempre - e con noi tutti gli italiani - il loro tributo alla sicurezza delle nostre comunità e alla difesa dei valori che incarnano la nostra Repubblica. Se, tuttavia, abbiamo garantito che per vent'anni l'Afghanistan non tornasse a essere un luogo sicuro per il terrorismo internazionale, non possiamo nasconderci il fallimento nell'attività di costruzione di istituzioni solide e realmente rappresentative dell'articolata società afghana. Su questo punto, quello cioè dell'*institution building*, siamo chiamati a riflessioni, che dovremo condurre sia nei contesti internazionali che a livello nazionale, relativamente ai nostri modelli di intervento e alla necessità di un approccio multidimensionale coerente, efficace e condiviso, di cui la dimensione militare è solo una delle componenti. L'esperienza afghana ci interroga, però, anche su quali conseguenze possono scaturire dalla crisi in atto e sugli impatti che questa potrà avere in un'area già di per sé fragile e che gioca un ruolo centrale negli equilibri geopolitici globali. In una prospettiva più generale, dobbiamo evitare che l'Afghanistan torni a essere un luogo sicuro per la *jihad* mondiale e i recenti attentati a Kabul, con il connesso significato propagandistico, possono essere strumentalmente presentati come una vittoria e una rinnovata affermazione delle capacità operative della galassia jihadista. Vi è il rischio, quindi, che il deterioramento del quadro di sicurezza si estenda a quelle regioni di elevato interesse strategico nazionale in cui siamo impegnati, quali il Sahel e l'Iraq. Chiaramente le condizioni di riferimento sono profondamente diverse: in Iraq - ad esempio - sta crescendo in maniera significativa la forza delle istituzioni e la NATO ha l'occasione di rilanciare le proprie capacità di *institution building*, mettendo immediatamente a sistema le criticità emerse nello scenario afghano. Sarà con questa visione di insieme, in particolare, che l'Italia, a valle di una ponderata e approfondita valutazione anche di quanto avvenuto oggi in Afghanistan, assumerà nel prossimo 2022 il comando della missione NATO in quel Paese. Nell'indicare le aree di interesse nazionale che potrebbero essere interessate dalle ricadute della crisi afghana ho prima citato il Sahel, regione che è sempre più centrale negli interessi di sicurezza europei e italiani e nella quale il nostro impegno è significativamente cresciuto. Anche qui dovremo portare le lezioni apprese dalla vicenda afghana in termini di modello di intervento e approccio a 360 gradi rispetto alle problematiche di quei Paesi. È evidente che il nostro Paese, così come l'Alleanza atlantica, deve trarre numerosi insegnamenti dall'esperienza afghana, per meglio identificare quali sono i suoi punti di forza, ma anche le sue debolezze, quale appunto la difficoltà a supportare un processo multinazionale di *nation building*, come quello che pretendeva lo scenario operativo afghano. L'epilogo afghano ha rilanciato la discussione in merito al ruolo della NATO e dell'Unione europea nello scenario globale. La NATO è stata e resta l'organizzazione di riferimento per la nostra sicurezza, che garantisce protezione e deterrenza rispetto all'evoluzione del quadro geostrategico mondiale e che, prima di essere alleanza militare, è innanzitutto alleanza di valori. Le democrazie liberali e il loro patrimonio di valori e diritti sono un modello da difendere, che, pur a valle dall'indispensabile processo di riflessione e di analisi sugli esiti dell'esperienza afghana, dovrà continuare a essere l'archetipo di riferimento del nostro peculiare apporto allo scenario di cooperazione e insieme di competizione del nuovo contesto globale. Il processo di revisione strategica NATO 2030, attualmente in corso, dovrà tenere in assoluta considerazione quanto avvenuto dal 2001 ad oggi, nello sviluppare il nuovo concetto strategico di una NATO bilanciata, ma soprattutto l'idea di alleanza del futuro e delle sue relazioni con le grandi organizzazioni internazionali, prima fra tutte l'Unione europea. L'Unione è chiamata ancora di più a definire coraggiosamente la propria autonomia strategica, in complementarietà con la NATO, ma valorizzando al massimo le peculiarità e gli strumenti che le sono propri, essendo l'organizzazione che più di tutte ha le capacità di intervenire con efficacia nella realizzazione di azioni proiettate allo sviluppo economico, culturale e sociale dei Paesi in cui siamo chiamati a operare. Il tema della difesa comune, oggetto della recentissima e autorevole sollecitazione del Presidente della Repubblica, è tornato centrale nella discussione politica europea, anche grazie all'azione propulsiva del nostro Paese. Iniziative concrete sono state avviate per promuovere una più forte integrazione nel settore, attraverso l'irrobustimento delle capacità, lo sviluppo di una più solida base industriale e l'adattamento dell'architettura istituzionale dell'UE, ma non basta: è necessario un salto di qualità, innanzitutto politico. Credo sia infatti ormai chiaro a tutti - la crisi afghana ce lo dimostra plasticamente - che siamo chiamati ad assumerci responsabilità sempre maggiori, nel quadro di quella che già oggi si chiama, non a caso, politica di sicurezza e difesa comune e che, attraverso la definizione della bussola strategica, dovrà finalmente trovare una sua direzione, insieme concreta e coraggiosa, per la quale la difesa europea vada perciò vista non esclusivamente come la risposta ad un'esigenza operativa, quanto piuttosto come un tassello fondamentale e necessario alla costruzione di un'Europa più pienamente politica, indispensabile per poter competere e agire sulla scena mondiale. Si tratta quindi di promuovere una maggiore assunzione di responsabilità da parte dell'Unione nel campo della difesa e della sicurezza, non in contrapposizione, ma anzi in piena sinergia con la NATO. Come ho in più occasioni sostenuto, la convinta promozione dello sviluppo e dell'acquisizione di capacità militari europee deve essere infatti assolutamente interpretata quale naturale e coerente azione di rafforzamento del pilastro europeo dell'Alleanza atlantica, a conferma dell'insolubilità del solido rapporto transatlantico e con l'obiettivo di consentire all'Europa di contribuire in maniera sostanziale ed efficace alla sicurezza e alla stabilità globale. Per fare ciò sono necessari un orizzonte politico e una visione comune: analisi delle minacce, definizione di un'agenda politica condivisa, costruzione di capacità militari comuni e, soprattutto, volontà di utilizzarle come Unione. Durante la riunione ministeriale UE di Lubiana della scorsa settimana abbiamo affrontato proprio il tema del ruolo che l'Unione vuole giocare nel contesto globale, partendo dalla lezione afghana, che deve essere di stimolo per rafforzarne il coraggio e il livello di ambizione. È evidente che, per entrambe le organizzazioni, una delle sfide riguarderà anche e soprattutto i processi decisionali. La nuova competizione globale richiede certamente rapidità ed efficienza: dovremo essere capaci, tutti noi, di rispondere a questa esigenza continuando a tutelare i principi e le forme delle democrazie liberali. Si tratta di una sfida certamente difficile, ma credo ineludibile, dentro i processi di revisione strategica delle organizzazioni internazionali di riferimento. Presidente, onorevoli senatrici e senatori, l'operato dei nostri militari, silenzioso e instancabile, merita il plauso e la gratitudine da parte dalla Nazione, per l'impegno al servizio dei valori della libertà e della democrazia in diverse regioni del pianeta, agendo con riconosciuta professionalità e sacrificio. L'evacuazione appena conclusa, il quotidiano impegno in patria e all'estero, il supporto nella lotta alla pandemia sono mirabili esempi di uno straordinario patrimonio umano di competenze e di conoscenza, sostenuto da irrinunciabili capacità tecnologiche, che dobbiamo preservare e sviluppare. L'esperienza afghana ci chiama alla responsabilità di plasmare una nuova architettura di difesa e sicurezza, incentrata sull'evoluzione e la fattiva collaborazione tra una NATO più moderna e un'Unione europea più forte, che considero, in tutta la loro portata, le sfide emergenti e il ruolo degli attori globali. L'Italia, anche attraverso un dibattito che sia all'altezza di questa sfida, deve continuare responsabilmente a fare la propria parte e lo farà. *(Applausi)*.

il merito di avere spianato la strada tra noi, oggi, a una riflessione seria, serena e sincera. serena e sincera. Lo meritano i più di 50 militari italiani caduti in Afghanistan affinché il loro sacrificio estremo non si riveli vano. Lo meritano i diplomatici italiani, i volontari e la straordinaria rete rappresentata qui in Parlamento che ha dato una prova straordinaria di abnegazione e di difesa degli interessi e dei valori della nostra patria. Colleghi, dicevo che è necessaria una riflessione seria - consentitemi un termine - e forse anche spregiudicata. Non basta la diplomazia in questo caso, soprattutto per noi parlamentari che non abbiamo dei doveri di siffatto tipo, ma è necessario guardare in faccia la realtà. in Iraq. Il presidente Bush decise l'invasione dell'Iraq e alla caduta di Saddam Hussein gli americani fecero seguire la decapitazione politica - ovviamente non sto parlando di quella fisica - di tutti i vertici sunniti dell'Iraq. Il risultato della vicenda e di questa scelta dell'Occidente fu che quindici anni dopo il califfato islamico dell'ISIS, insediato tra l'Iraq e la Siria, fu in gran parte figlio non solo di quei fuoriusciti di Al Qaeda e dei terroristi, ma anche dei vertici sunniti che costituirono in Iraq e in Siria la base di riferimento politico-istituzionale del califfato che si sarebbe andato a insediare. Un errore capitale dell'Occidente è stato la causa di uno dei fatti più pericolosi per l'Occidente, e cioè la nascita del califfato dell'ISIS.

si è trovato a consegnare armamenti di primo piano e di nuova generazione ai talebani, questo non può essere una casualità. Questa è la conseguenza di governanti corrotti che l'Occidente ha appoggiato a piene mani e che sono stati i primi a scappare

che i padroni e i signori della guerra in Afghanistan in questi anni - ad esempio - non hanno limitato la coltivazione di droga, ma l'hanno incentivata. Dopo l'occupazione occidentale abbiamo consentito che ci fossero governanti di uno Stato narcotrafficante e oggi ci meravigliamo che non abbiano combattuto. Questi governanti sono stati i primi a scappare e sono stati i primi ad avere usufruito in larga misura degli aiuti che noi abbiamo dato loro istituendo una statualità che speravamo potesse resistere. Naturalmente, quando dico noi, parlo dell'Occidente e non mi riferisco al Governo italiano. Noi siamo una piccola parte di questo ingranaggio, ma oggi dobbiamo riflettere sugli errori dell'Occidente. Colleghi, mi chiedo se davanti a fatti di questo tipo abbia senso il dibattito che quest'estate è fiorito sul tema dell'esportazione della democrazia. Guardiamoci in faccia: se per esportazione della democrazia intendiamo l'esportazione di modelli parlamentari occidentali, in realtà come l'Afghanistan o anche come la Libia, allora è chiaro che non possiamo esportare la democrazia. Se, invece, per esportazione di democrazia intendiamo - come io intendo un reticolato di diritti indisponibili che la dignità dell'uomo afferma in qualsiasi parte del mondo

della nostra tradizione e della nostra cultura. Ma non possiamo rinunciare a pensare che questa non sia un'aspirazione umana che valga per l'Afghanistan come per qualsiasi area desolata e isolata del mondo. mondo. Qui non si tratta di fare penitenza perché abbiamo cercato di esportare la democrazia, perché la parte delle relazioni di Di Maio e di Guerini che - secondo me - è più convincente e motiva il sacrificio dei nostri militari - questo sì - è che siamo riusciti finalmente a esportare diritti che hanno consentito al popolo afghano di andare a votare, di rispettare la dignità delle donne, di vedere le donne nelle posizioni di guida della società, di vedere i minori andare a scuola. Di Maio ha rilevato

dobbiamo riconoscere che quello che è successo in Afghanistan, a Kabul, in quei terribili giorni di agosto, è uno spartiacque a vent'anni dall'11 settembre. Non è un qualcosa a cui dobbiamo reagire con una sorta di formalismo del quotidiano. Colleghi, l'Occidente ha un senso? E ancora, che cos'è l'Occidente? Sono interrogativi da cui un Parlamento come questo, un Parlamento di un Paese come l'Italia, che nel 1948 ha scelto l'Occidente, che orgogliosamente rivendica l'amicizia con gli Stati Uniti proprio perché si sente parte di quest'anima occidentale, deve fare una riflessione al riguardo. Credo a questo punto - e mi avvio alla conclusione - che la riflessione vera da fare sul tema dell'Occidente è che, se continuiamo a ritenerci occidentali, affidando agli Stati Uniti d'America la possibilità di essere il *dominus* e anche in qualche modo l'unico punto di riferimento vero di questo Occidente, temo che la risposta l'abbiamo avuta a Kabul. Temo che questo tipo di Occidente rischi di non esistere più, perché non possiamo non vedere che la politica americana è profondamente cambiata. È cambiata con Trump? Qualcuno si illudeva che fosse cambiata con Trump.

vero che la linea di continuità parte da Obama, passa attraverso Trump, arriva a Biden e, sotto il profilo della solidarietà occidentale, c'è una continuità che pone noi, europei e italiani, davanti alle nostre responsabilità. Crediamo che l'Occidente abbia una funzione? Se crediamo a questo, non aspettiamoci più niente dagli Stati Uniti d'America che non possiamo fare noi. Non è più il tempo delle deleghe alla superpotenza e sapete perché? La superpotenza non c'è più, perché oggi abbiamo una serie di attori che entrano nello scenario - ad esempio del dopo Afghanistan - che mettono drammaticamente ciascuno davanti alle responsabilità. Noi stiamo aprendo gli occhi oggi per le immagini terribili degli aerei che decollano e della gente attaccata alle loro ruote. Ma dovevamo accorgercene prima, colleghi, perché quando gli attori europei sono andati avanti in ordine sparso, in scenari ben più difficili dell'Afghanistan - penso alla Libia - il risultato è stato quello che vediamo; gli attori libici sono il Qatar, la Turchia e la Russia; Italia e Francia contano poco più di zero. Illudiamoci che non sia così, ma tra di noi poi, in privato, sappiamo che è così. Ed è così perché hanno deciso di giocare delle partite diverse su tavoli diversi. Il risultato è che entrambe le partite

se non c'è un polmone unico di politica estera. A cosa volete che servano 10.000 uomini messi assieme nella politica di difesa? Noi dobbiamo riportare al centro del villaggio - come direbbe qualcuno - il seguente tema: se vogliamo che l'Occidente esista, dobbiamo fare la nostra parte e tutti i signori protagonisti della politica europea internazionale

piani diversi. Oggi invece devono venire assieme perché, se parliamo di Afghanistan, sappiamo che la politica di difesa è strumento di una scelta di politica estera e i due

e avere il coraggio di dire che noi concentriamo gli sforzi nelle aree in cui geopoliticamente c'è più interesse per l'Europa e per il nostro Paese. Penso che, detto ciò, detto ciò, va rilevato che noi certamente abbiamo sofferto per questo epilogo, ma ci auguriamo che oggi

che questi cinque punti vengano rispettati. Sono contento che nessuno lo abbia proposto in questa sede. Qualcuno a volte butta il cuore oltre l'ostacolo, ma credo che sarebbe veramente un tradimento anche di quei concetti di serietà che siamo impegnati ad affermare.

penso che sia vero soltanto in parte: siamo alla fine di una stagione, alla fine di quello che in tanti abbiamo chiamato il secolo americano. Chi come me è convintamente filoatlantico, grande sostenitore dell'amicizia con gli Stati Uniti e convinto difensore dei valori che la nostra Alleanza ha sempre portato avanti, soffre per questo giudizio. E nell'affermarlo, purtroppo, è il momento di dire con chiarezza ad alcuni antiamericani del giorno dopo, che hanno approfittato per alcune analisi a mio giudizio profondamente superficiali, che non è vero che gli Stati Uniti d'America hanno perso questa guerra, gli Stati Uniti d'America hanno perso questa guerra, bensì l'hanno vinta. Gli Stati Uniti d'America hanno perso insieme a noi il dopoguerra, ma negli obiettivi militari di distruzione degli attentatori e dell'organizzazione terroristica gli Stati Uniti hanno ottenuto un risultato. A chi dice che dopo l'11 settembre non si doveva intervenire militarmente vorrei ricordare dove eravamo noi, l'11 settembre. Pensavate forse che fosse possibile uno scambio di note diplomatiche, dopo che quelli avevano buttato giù le torri gemelle, colpito il Pentagono e cercato di colpire la Casa bianca? È evidente che la reazione militare dovesse essere la reazione. Gli americani la guerra l'hanno vinta e a chi ancora oggi sui giornali italiani qualche ora fa scriveva che Osama Bin Laden è il vero vincitore di questa guerra dei vent'anni, vogliamo ribadire, con molta umiltà, da dove festeggia Osama Bin Laden la sua presunta vittoria? Dal fondo del mare dov'è sepolto, dopo che militari americani dieci anni fa lo hanno giustiziato come era doveroso fare. A chi ancora oggi - l'ha detto perfettamente il ministro Guerini, che ringrazio - dice che si sono persi la guerra e il dopoguerra perché i nostri erano male organizzati, non è stato un problema di cattiva formazione. Onore alle donne e agli uomini dell'alleanza, onore alle donne e agli uomini italiani e non soltanto italiani che hanno formato gli afghani. Tutti noi siamo stati ad Herat insieme a loro e abbiamo visto la loro professionalità. Si è perso il dopoguerra per la corruzione dei signori della guerra afghana che scappano con 169 milioni di dollari da un elicottero lasciando dei contanti sulla pista; si è voluto e non si è stati capaci di costruire un'entità statale - perché non era facile - e perché non si sono avuti la forza ed il coraggio di immaginare una grande sfida di natura culturale ed educativa vincente. È accaduta - vedo la senatrice Pinotti, che allora svolgeva il ruolo che oggi è del ministro Guerini la stessa identica cosa, pur in circostanze profondamente diverse, quando l'esercito iracheno ben formato e ben equipaggiato ha scelto di non combattere il 10 giugno del 2014 a Mosul. Ricordatevi quella vicenda: allora l'esercito iracheno scappò davanti a quello che stava costituendosi come Stato islamico, Daesh, e in quella fuga vergognosa nacque una organizzazione criminale e terroristica che ha colpito non soltanto in quel territorio, ma che per un effetto emulativo sul quale proverò a tornare ha poi colpito l'Europa. In quella vicenda,

a chi stava combattendo sul territorio contro gli estremisti islamici. In quella vicenda fu decisivo il ruolo delle donne curde, che combatterono in prima linea per la libertà non solo del loro territorio, poi abbandonato di nuovo dall'alleanza, ma anche di tutte e tutti noi.

era il messaggio di Trump e spiace dire che è stato recepito anche dalla corrente amministrazione americana. Lo dico con la morte nel cuore e con stima e amicizia nei confronti dei *leader* americani. Lo dico ricordando le parole di Joe Biden di qualche settimana fa. Alla fine della battaglia sui vaccini, vaccini, sottolineando il successo degli americani e dell'organizzazione americana in tema di vaccinazione, disse: soprattutto questa vicenda è la prova che la democrazia funziona, che le democrazie funzionano e che, ancora una volta, l'America torna a guidare il mondo non con l'esempio della nostra potenza, ma con la potenza del nostro esempio. Noi siamo gli Stati Uniti d'America; noi siamo pronti come mai prima. Abbiamo gli strumenti e le risorse per salvare vite a casa nostra e nel resto del mondo. Questo siamo noi e questo facciamo noi perché non c'è alcuna Nazione come noi sulla terra. Queste sono le parole di Joe Biden quando spiega il successo della campagna vaccinale. Le avrei volute sentire, ma così non è stato, anche sulla vicenda afgana. È un dato di fatto: cambierà molto nella politica americana e avremo modo di riparlarne. Questa è la discussione da fare di politica estera, con la Cina che oggi è il principale soggetto dell'area e si accinge a guidare il secolo asiatico, ma che è anche la prima interessata a evitare che l'Afghanistan diventi un luogo di terrore. La Cina è oggi sul breve periodo la vincente, ma sul medio periodo avrà da gestire una serie di preoccupazioni diverse. A tal proposito, non va sottovalutato il rapporto tra Cina e Russia,

nel mondo sunnita, in quanto potrebbero tornare a dialogare i mondi sunniti che non si parlavano e ciò potrebbe provocare una diversa reazione anche da parte degli indiani. Infatti, non dimentichiamo che Pakistan e India in questo periodo hanno avuto molti elementi di tensione. Per quello che ci riguarda, signora Presidente, c'è una vittima sul campo. Le prime vittime, naturalmente, sono le persone che hanno perso la vita, a cominciare da quelle dell'aeroporto;

ma anche di diversità di toni diplomatici. C'è il problema della NATO, che è grande come una casa. La NATO è una vittima collaterale di questa vicenda. Quando Emmanuel Macron parlava di morte cerebrale della NATO, tutti a dire che non è cerebrale. È morte.

gestendo. È evidente che, a quel punto, se non c'è la NATO ci deve essere, come minimo, l'esercito europeo. Delle due l'una: o la NATO si mette a funzionare, oppure abbiamo bisogno di una reazione europea. Anche perché altro che comportamenti distensivi dei talebani! talebani hanno ammazzato un premio Pulitzer a luglio e hanno ucciso comici, musicisti e donne. Ma quali comportamenti distensivi? Ha ragione il ministro Di Maio a dire di giudicarli sui fatti, ma i fatti hanno già parlato.

Noi pensiamo che la questione del terrorismo riguardi l'emulazione di fenomeni come quelli verificatisi nel 2014-2015 quando, dopo quanto accaduto in Siria, i lupi solitari e le persone nelle *banlieu* hanno iniziato a farsi esplodere in Europa. Questo è il dramma e su questo bene ha fatto il Governo a convocare il G20 e bene hanno fatto i Ministri a lavorare in questa direzione; lasciatemi dire, però, che c'è una grande e gigantesca battaglia educativa e culturale che tutti insieme dovremo vincere e che non è facile da giocare nei prossimi anni.

di essere venuti questa mattina qui in Senato, anche se avrei voluto il dibattito parlamentare quando fu deciso

ma dalle azioni i talebani e quello che sarà il Governo dell'Afghanistan. Signor Ministro - questo peraltro vale anche per noi, vale sempre e dovrebbe valere per tutti, anche per il Governo italiano - restando a quello che lei dice, credo che siamo messi veramente male. Ho infatti il dispiacere di annunziare che cinque minuti fa, mentre parlava il collega Casini, mi ha chiamato da Kabul il giornalista Micalessin

la lunga sequela di cifre, di euro che verranno dati per la moralmente doverosa ricostruzione e per gli aiuti umanitari, ma guai se queste risorse dovessero arrivare attraverso il Governo afghano, attraverso i talebani, perché vogliamo sapere fino all'ultimo centesimo a chi andranno e attraverso chi. Sia ben chiaro. Non facciamoci prendere dalla solita faciloneria umanitaria, che deve essere invece reale e condivisa,

furono coloro che determinarono l'intervento. Infatti, se il Governo afghano di allora avesse risposto all'*ultimatum* occidentale, degli Stati Uniti in particolare, che chiedeva di consegnare gli autori e il capo degli autori degli attentati dell'11 settembre, non ci sarebbe stato l'intervento in Afghanistan che, sia ben chiaro, fu doveroso e oggi io lo rivendico, anche se non ero in maggioranza. Lo ha rivendicato benissimo il Ministro della difesa, quindi è un segno di quella opposizione patriottica che è tipica di Fratelli d'Italia (dare a Cesare quel che è di Cesare). Quell'intervento fu motivato dalla necessità di impedire che il terrorismo fosse vicino a casa nostra;

che si era manifestato non solo con l'attentato alle Torri gemelle, ma con gli assalti alle ambasciate, con bombardamenti e con le bombe in mezzo mondo. Questo bisogna ricordarlo

È stata un fallimento politico innanzitutto perché c'era chi andava lì per combattere i talebani e c'era chi andava lì solo per ricostruire. Per anni anche l'Italia, non dopo una certa data, creduto che i nostri soldati fossero lì a distribuire acqua minerale. Non era così: eravamo lì per contrastare la ferocia dei talebani ed è stato fatto con un grave sacrificio umano. È toccato a me, come sa la senatrice Pinotti, il periodo più duro, quando sulle mie spalle ho portato le bare di tanti, troppi, giovani che oggi vanno ricordati non solo con le parole, ma con la testimonianza dell'attenzione che - lo dico sottovoce - questo Governo ha mancato nel momento del rientro, perché nessuno è andato ad accogliere la Folgore che tornava da Kabul, neanche uno straccio di Sottosegretario *(Applausi)*. Ripeto, neanche uno straccio di Sottosegretario.

una fase in cui l'Europa dovrà avere un peso diverso, perché diverso è il ruolo della NATO, che è già cambiato dopo il 2011: non c'è più stata una sola missione internazionale, dopo quella in Libia del 2011. un Europa attrezzata. Non è questa Europa, per questo noi parliamo di confederazione europea, a cui siano riservati dei compiti veri di difesa, di politica estera, certo di gestione del fisco e della moneta, certo delle grandi questioni anche di immigrazione, ma che per il resto sia rispettosa delle

prioritaria nell'agenda politica europea. Noi ci aspettiamo che contestualmente una politica per una difesa comune

È questa l'ambizione di un'Europa seria, di un'Europa che ci piacerebbe, che fa le cose importanti invece di accodarsi soltanto alle decisioni degli americani, che hanno sbagliato non solo

Il ritiro andava commisurato alle condizioni, non ai tempi. Abbiamo fatto un regalo enorme ai talebani. Il tempo sta per

Io sono stato a Bala Murghab, sono stato a Farah, certo anche ad Herat e a Kabul, ma in quegli avamposti ho visto il valore dei nostri militari. Un avamposto grande come questa sala, bombardato ogni giorno dai mortai. Erano lì perché? Me lo chiedo anche oggi e me ne sono fatto una ragione: per combattere contro il terrorismo, ancor prima che per portare o introdurre forme di democrazia che quel popolo non voleva. Erano lì per testimoniare la volontà del popolo italiano di essere partecipe e protagonista di un'azione di pace che non può avvenire senza Forze armate adeguate e sostenute, anche economicamente, dai Governi che troppe volte fanno orecchie da mercante.

Concordo con quanto ci ha detto il Ministro oggi e ci aveva detto anche nelle audizioni, in risposta alla domanda se non fossimo potuti rimanere noi senza gli americani. No, una missione così complessa, con quel tipo di organizzazione, non poteva prevedere distinzioni in quel momento.

Davvero c'è da chiedersi perché in quel momento si dialoga con i talebani e non prima, per esempio, quando avevamo una posizione di forza ben diversa, capendo che comunque vi era una forza presente e si poteva aprire, ad esempio dopo l'uccisione di Osama Bin Laden? di farlo in quel momento, quando già si dice che ci si sarebbe ritirati, mettendoci quindi in una posizione di grande debolezza.

negativi che ho ascoltato questa mattina e nelle relazioni dei Ministri, alcuni più delicati, altri più diretti, ma fino a quel momento era il Governo legittimo, pur con tutte le debolezze del caso. Non ci

non ha combattuto, sicuramente anche perché il Governo non ha saputo creare quella coesione e quella motivazione che ci devono essere per combattere. Ricordo i peshmerga curdi, addestrati dalle nostre Forze, come hanno combattuto contro l'ISIS. Il popolo afghano

Evidentemente si sono trovati scoperti e credo che anche la trattativa aperta con i talebani senza il Governo legittimo sia stato un elemento che li ha fatti sentire scoperti. Mi associo ai ringraziamenti al corpo diplomatico, alle nostre Forze armate straordinarie e all'*intelligence* per quanto abbiamo fatto per l'evacuazione, non soltanto per i numeri che oggi avete dato, ma anche per le modalità. Ho sentito delle testimonianze di giornalisti italiani, che sono rimasti colpiti per come i nostri militari non solo facevano salire le persone sugli aerei, ma per come li facevano sedere ai loro posti, come a ciascuno davano il proprio pranzo, cioè con un'attenzione e una gentilezza che ha veramente colpito i giornalisti che conoscevano meno l'operato delle nostre

la discussione che è stata fatta in Europa, sia per quello che riguarda il piano nazionale. Positive le condizioni poste in Europa, quindi distinguiamo: se

anche il G20, perché è un *forum* che stiamo presiedendo e che può diventare un'occasione importante. Credo che, fra tutto quello che ci siamo detti, il punto centrale l'ha toccato anche il senatore Casini: il tema dei diritti. Penso sia inutile adesso aprire la discussione su come si costruisce una democrazia. Non c'è dubbio che lo sforzo anche dei nostri militari e dei

Non c'è dubbio che non è da ora che gli Stati Uniti dicono: sul vostro quadrante, sul Mediterraneo e sul Medioriente, che cosa pensate si debba fare? Voi fate e noi comunque vi aiutiamo. L'investimento sul fatto che noi dobbiamo assumerci le nostre responsabilità non è da ora, ma dopo un avvenimento come questo in Afghanistan non possiamo più fare "passetti" dobbiamo veramente dare una svolta sul tema della difesa europea, che non è in contrasto con la NATO. Poi discuteremo se la NATO è davvero morta oppure no e quale deve essere il concetto strategico. Ma fino ad ora rappresenta un'alleanza strategica fatta anche di valori, quindi starei attenta a buttare via tutto. Io penso che la NATO diventa più forte, più autorevole, più competente e più capace di intervenire nel mondo se, oltre al punto di vista degli Stati Uniti (che c'è fortissimamente), c'è anche una prospettiva che diventa forte se è un punto di vista europeo e non solo delle singole Nazioni. La costruzione di una difesa europea, come avete detto non è questione tecnica: tecnicamente ci si mette pochissimo a farla, non è questo il problema; il problema è politico e scegliere che l'Europa si muova nel mondo con una propria direzione e scelte di politica estera che fanno capire che cosa vuole essere l'Europa nel mondo. Ripeto, tecnicamente non è difficile e si può fare. mi chiedo: se non ora, quando? Questo è il momento.

conoscendomi, sapete benissimo che non amo fare politica con il retrovisore, guardando indietro; normalmente cerco di farla guardando avanti. In questa occasione, però, ci sono due o tre punti fondamentali che mi sfuggono e su cui chiederei delle risposte più chiare. chiare. Ho letto, riletto e conosco quasi a memoria lo scarno testo del cosiddetto accordo di Doha: quattro paginette. L'ho letto e riletto. Ho letto che, da una parte, c'erano gli Stati Uniti e «its allies», genericamente parlando. Non so a chi si riferiscano, se alla Nato a noi. Comunque, da una parte, c'erano, appunto, Khalilzad e Pompeo e, dall'altra, i talebani. È un segreto di Stato sapere chi c'era per i talebani? talebani? A parte il signor Baradar, che peraltro è riconoscibile, chi rappresentava il signor Baradar?

almeno informati? In questo testo, la NATO non viene neanche citata. Eppure, sappiamo bene che si era in Afghanistan con una missione NATO che si chiamava all'epoca ISAF, alla quale noi partecipavamo, peraltro con un via libera del Consiglio di sicurezza. Se capisco bene, anzi lo capisco benissimo, la NATO non è neanche citata. Si citano gli americani «and its allies»: mi piacerebbe sapere a chi si riferiscono.

un altare! Perché è importante sapere chi c'era e chi rappresentava chi a questo tavolo?

prima questione. La seconda è la seguente. Sempre leggendo e rileggendo questo accordo, i diritti umani delle donne o dei bambini non sono neanche citati, neanche evocati, neanche evocati, neanche per ipocrisia. Non ci sono. L'unica cosa che Pompeo e Khalilzad chiedono ai talebani, genericamente parlando, è di rompere i rapporti con la parte jihadista.

o USA, come preferite) è strabiliante. Possibile che, in un territorio controllato da truppe occidentali, non ci si accorge che è nato questo ISIS Khorasan,

Sono contenta che l'Europa abbia messo i paletti anche sui diritti umani, ma state attenti perché nell'accordo che vorremmo monitorare non sono citati neanche lontanamente.

Draghi e Xi Jinping) abbia luogo, perché questo è l'unico modo per riuscire a capire se almeno una qualche sintonia per evitare la guerra civile sia ancora possibile. Infine, devo dire che condivido, ministro Guerini e ministro Di Maio, quanto avete detto sulla difesa. Guardate che, se non c'è una politica estera, della politica di difesa non ce ne facciamo niente, se non per l'emergenza ambientale: se c'è un alluvione, chiamiamo i nostri 5.000 militari. Ma per tutti gli altri casi che abbiano implicazioni, senza politica estera non

Temo che sarà difficile mantenere questa posizione, perché è evidente che Russia, Cina, certamente Turchia e altri Paesi arabi li riconosceranno. Non siamo quindi prego però di tenere questa posizione e di appoggiare a Ginevra l'istituzione di una commissione indipendente di monitoraggio, in modo che questa nostra uscita non

Signor Presidente, signori Ministri, colleghi senatori, chiariamo subito un concetto: l'emergenza è umanitaria, ma la crisi è politica. Ridurre una gigantesca, colossale crisi politica all'emergenza umanitaria, che pure ne discende, è un segno di insipienza ed è forse il più evidente segno dell'avvenuto tramonto dell'Occidente. Siamo arrivati a questo punto non a causa di politiche sbagliate, ma a causa di una drammatica mancanza di politica, di senso politico. È mancato il senso politico ai Paesi della della NATO, in generale, e agli Stati Uniti in particolare quando hanno pensato di organizzare un cambio di regime non dal basso, non coinvolgendo i diversi *clan*, le diverse etnie, le diverse tribù, non coinvolgendo i Paesi dell'area, - come era stato fatto, sbagliando, in Iran prima della rivoluzione di Khomeini, in Iraq dopo la caduta di Saddam, in Somalia alla fine dell'operazione Restore hope - calando dall'alto il potere su una serie di lacchè lacchè locali che naturalmente, alla prima difficoltà, si sono dissolti come neve al sole. Il problema ha radici antiche a mio avviso. Dopo la carneficina della Prima guerra mondiale, sulla spinta dell'idealismo della presidenza americana di Woodrow Wilson, con il patto Briand-Kellogg, la comunità internazionale si diede un obiettivo ambizioso: mettere al bando la guerra. Da allora cominciò un processo culturale che ha attraversato tutte le società occidentali e che ha portato a sostituire, di fatto, la logica politica con quella umanitaria. Il problema è che la logica umanitaria non giustifica i morti in battaglia. Assistiamo quindi a un paradosso, per cui la potenza globale per eccellenza, gli Stati Uniti, non ha più la forza morale di considerare la morte come un evento naturale nell'orizzonte di chi sceglie liberamente il mestiere delle armi. Tutto il resto ne consegue: possiamo anche ribattezzare «pace» la guerra, ipocritamente, come siamo abituati a fare, possiamo anche appaltare ai privati la guerra, per non avere la contabilità dei morti, possiamo anche - come facciamo anche noi italiani nella parata del 2 giugno nascondere le nostre Forze armate, dietro funzioni e figure sempre più eminentemente civili, ma questo non ci mette in grado di affrontare i problemi, quando essi fatalmente si manifestano. Anche aver ridotto il senso della guerra in Afghanistan alla questione dei diritti umani e della democrazia, giusta in astratto, è stato un elemento di debolezza. Considero esportabile la democrazia, ma in tutta non nei tempi che la comunità internazionale si era data. Quindi siamo andati incontro ad un fallimento annunciato ed è stato un peccato, perché è vero che la società afghana non si è democratizzata in questi vent'anni, ma è altrettanto vero che si è evoluta enormemente, il PIL è triplicato, la mortalità infantile si è dimezzata, l'alfabetizzazione è aumentata di oltre il 50 per cento. Sono dei successi, considerati come sconfitte, perché c'eravamo dati un obiettivo sbagliato. Anche ridurre ora tutto alla questione umanitaria è pericoloso e scivoloso: quand'anche riuscissimo - e non ci riusciremo - ad espatriare tutti gli afghani che vogliono abbandonare il loro Paese, con ciò dimostrando che un progresso c'è stato,

giocoforza - della logica umanitaria e aderire ad una logica politica. Bisogna fare politica, con quella logica politica che gli Stati Uniti stanno dimostrando di non riuscire più a sostenere e che noi italiani e noi europei non abbiamo mai avuto. Colleghi, diciamoci la verità: non abbiamo mai avuto una politica estera e lo dico con rispetto per il ministro Di Maio e per i tanti che l'hanno preceduto, perché non è possibile avere una politica estera senza una politica della sicurezza. Abbiamo delegato la nostra politica della sicurezza agli Stati Uniti ed ora che gli Stati Uniti - con Biden, ma in linea con Trump - si ritirano dal mondo, siamo soli, indifesi e incapaci di politica. Il problema si risolve con una forte iniezione di realismo e di politica. La questione della difesa comune europea è l'obiettivo: occorre ripartire dal 1954, dalla data famigerata, in cui il Parlamento francese bocciò quel progetto e riattualizzarlo, ma per farlo bisogna uscire dalla logica umanitaria e avere senso politico. Colleghi, non è una possibilità, ma è una necessità imposta dal disarmo americano e dall'incombere di grandi potenze, come la Cina di Xi Jinping e, ahimè, la Turchia di Erdogan. Signor Presidente, membri del Governo, colleghe e colleghi, internazionale, a fronte di una crisi geopolitica così delicata, complessa ed importante, che investe anche il nostro Paese, ci aspettavamo che questa informativa in Assemblea fosse di assoluta priorità. Peccato per questa inspiegabile lungaggine e per questo ritardo! Si potrebbe dire: meglio tardi che mai, ma non intendo

Non si può che partire da un punto fondamentale: il degenerare della situazione in Afghanistan dimostra che la democrazia non è esportabile, laddove non supportata da dovuti presupposti e laddove non vi siano altri interessi predominanti. Pensare di cambiare o imporre la cultura altrui è inaccettabile, soprattutto quando non sono chiari gli obiettivi di una simile politica, poiché ogni popolo ha un suo processo storico e culturale. Non dobbiamo farci tentare farci tentare dal desiderio di esportare la democrazia, ma sarebbe meglio concentrarsi sulla tutela dei diritti umani a livello globale, i quali non hanno confini nazionali. Ciò deve avvenire solamente attraverso azioni mirate e con la diplomazia, insieme a una lotta decisa contro il terrorismo internazionale. Questo è il momento ideale per dimostrarlo. La politica estera non si basa esclusivamente sull'ideologia politica dei singoli partiti, ma sulla diplomazia multilaterale o sui soli interessi di ogni singola azione poiché la politica stessa non si fonda su sensazioni o prime impressioni, ma sul realismo e, cioè, la capacità di leggere e interpretare le situazioni reali per come esse si presentano per arrivare a una soluzione di qualità. È questa capacità di coesione organizzativa che oggi manca all'Unione europea in un mondo che ormai già mostra gli effetti della globalizzazione anche dal punto di vista geopolitico. Non possiamo rischiare che l'Europa resti ai margini della politica estera o, peggio ancora, che subisca le decisioni di altre potenze mondiali. Ora ci troviamo ad affrontare le conseguenze della crisi. Dovremo tutelare i veri profughi, come contemplato anche dalle linee guida della nostra politica sull'immigrazione, attraverso uno sforzo comune condiviso da tutti i Paesi dell'Unione europea, senza dimenticare che dobbiamo trovare un'identità e una visione comunitaria in politica estera e non solo per combattere terrorismo e garantire la libertà e i diritti conquistati. È evidente che l'Italia da sola non possa accogliere centinaia di migliaia di profughi sia per limiti strutturali, sia per la necessaria cautela per evitare i rischi imminenti di infiltrazioni terroristiche.

Il rapido disimpegno dell'Occidente in Afghanistan e la contestuale ascesa dei talebani non può renderci ciechi e indifferenti innanzi alle scene cui abbiamo assistito. È, infatti, intollerabile limitarsi ad assistere a manifeste violazioni dei diritti umani della *rule of law*, unitamente a tragiche scene di un'imminente crisi umanitaria in corso. Tutto ciò non può che essere fonte di imprevedibili rischi globali legati a una situazione di assoluta instabilità e incertezza, in aggiunta a quelle libica, siriana e libanese. Il Parlamento deve essere il luogo di dialogo e discussione competente in quanto casa della democrazia. Ciò deve avvenire sia nelle scelte strategiche e tutele dei veri profughi, sia nella tutela del diritto del popolo italiano a vivere al sicuro dal rischio di immigrazione incontrollata e soprattutto di potenziali terroristi. Mai come oggi in questa sede serve una visione lucida dell'effettiva evoluzione dello scenario della crisi umanitaria e geopolitica affinché si possa arrivare a una condivisione di responsabilità tra tutti i Paesi coinvolti abbracciando due specifiche linee direttrici: la tutela dei diritti umani e la tutela della sicurezza internazionale. Esprimo, infine, un sentito ringraziamento alle nostre donne e ai nostri uomini che sono stati impegnati in Afghanistan. Penso a militari, poliziotti e civili che hanno svolto un immenso lavoro in quello che si è rivelato uno scenario estremamente complicato nello scacchiere globale. Un commosso pensiero va a chi è caduto per servire il nostro Paese *(Applausi)* a cui si unisce un sentito abbraccio ai familiari. Un altro importante ringraziamento va anche alle migliaia di afghani che hanno lavorato fianco a fianco con il contingente italiano: è stato confortante, nell'immagine della tragedia, vedere lo straordinario lavoro della nostra rete diplomatica nell'evacuare quelle persone. Sapere che il nostro Paese può regalare una seconda vita a chi ci è stato accanto nel corso di questi vent'anni

quanto sta accadendo in Afghanistan ci chiama in causa come donne e uomini. Le immagini strazianti dei profughi non possono lasciarci indifferenti: sono le sue parole, ministro Di Maio, e sono anche le mie. Ministro Di Maio, questo è esattamente il primo dei miei e dei nostri pensieri. A Kabul e in Afghanistan ci sono ancora moltissimi nostri collaboratori e le loro famiglie: donne, uomini, bambini - molti bambini che si nascondono o hanno tentato la fuga attraverso il Pakistan. Dopo gli attentati all'aeroporto di Kabul e la chiusura, sono rimasti soli. Giungono notizie di rastrellamenti casa per casa e di sicuro essi vivono in un terrore costante e per loro ogni secondo scandito dall'orologio pesa come un macigno. Dobbiamo portarli in salvo. Allo stesso modo, giornalisti e attivisti vengono arrestati proprio mentre stiamo discutendo. In questi giorni terribili ho avuto modo di interloquire con alcuni di loro, con personalità afghane, intellettuali, cittadini e attivisti riparati all'estero, ma che hanno le loro famiglie in Afghanistan, e hanno riconosciuto a lei, Ministro, e al nostro Paese una forza e una determinazione nelle operazioni di evacuazione che altri Paesi non hanno dimostrato. Lo posso confermare poiché anche io sono stato in quelle tragiche ore in strettissimo contatto con la Farnesina. Doppio è quindi il pregio del nostro Paese: il primo è umanitario, il secondo è aver acquisito, durante i recenti Governi grazie al lavoro del *premier* Conte, prima, di Draghi che ne ha raccolto i risultati e del suo lavoro, ministro Di Maio - una credibilità in Europa e nei rapporti internazionali che ora è evidente a tutti. La testimonianza è la sua missione in Uzbekistan, Tagikistan, Qatar e Pakistan; è il rapporto soprattutto con i suoi omologhi di Francia e Germania. Ora serve, per prima cosa, che l'Unione europea si muova unitariamente: un conto è valutare ed eventualmente agire nei confronti della diplomazia coi talebani, nonché in eventuali scelte, a mio avviso necessarie, logistiche e operative di assistenza, soprattutto negli aeroporti afghani, come Paese Italia; altro conto è farlo come Unione europea. Saremmo veramente una potenza. Ciò oggi è possibile proprio perché l'Europa, nella sua storia recente, in questo dramma afghano ha risvegliato una coscienza individuale e collettiva mai avuta prima. È un momento storico in cui veramente possiamo lavorare insieme. Secondo punto: anche con il dialogo internazionale nell'ambito del G20 dovrebbe essere l'Unione europea a parlare, o almeno una parte di essa estremamente rappresentativa. evidente a tutti, anche ai più critici e ai riottosi, che è inevitabile un dialogo con Cina, Russia e Turchia. Sono coloro che possono fare la differenza nella gestione della crisi. Non parlo degli Stati Uniti, ovviamente inclusi, ma che al momento non sembrano avere posizioni chiare in merito. Ministri, colleghi, Presidente, questa è una grandissima occasione, storica, per dimostrare a noi stessi e ai popoli europei che, in questo contesto internazionale, insieme possiamo essere un soggetto forte e pesante sugli equilibri geopolitici. È l'occasione di una nemesi e catarsi per tutta l'Europa. Questa è un'occasione per dimostrare e realizzare davanti al mondo che il nostro Paese è diplomaticamente e strategicamente ineludibile nelle crisi internazionali, soprattutto nei confronti di Cina, Turchia e Russia. Cito il presidente Mattarella, è stato netto su questa vicenda dicendo che quanto è successo nella guerra in Siria ha reso evidente la scarsa capacità dell'Unione europea di agire unitariamente, è invece indispensabile assicurare gli strumenti reali, efficaci e concreti di politica estera e di difesa comuni. Questi strumenti esistono e possono essere usati dall'Europa in contesto internazionale. Mi riferisco alla direttiva sulla protezione temporanea n. 55 del 2001 della Comunità europea sullo *status* di protezione di gruppo, che potrebbe essere applicata proprio per il caso Afghanistan, creando visti per tutti e corridoi umanitari. È un'opzione da portare in ambito internazionale con la forza dell'Europa. È l'occasione di salvare, signori, centinaia o migliaia di afghani che ci hanno aiutato, che sono stati nostri collaboratori, traduttori, impiegati e che sono perseguitati e profughi a causa nostra e della NATO e non possiamo fallire.

ai tantissimi rifugiati. Ciò non perché dobbiamo paventare chissà quale fuga, ma sappiamo perfettamente che dovremo saper gestire seriamente la questione dei rifugiati e qui arrivo al punto.

Qui abbiamo il problema. L'Italia si sta muovendo bene, ma c'è il tema di muoversi davvero in modo condiviso come Unione europea e devo dire che le prime riunioni dei Ministri dell'interno dell'Unione europea non sono andate proprio nella giusta direzione. È questo il problema e noi e noi dobbiamo saperlo perché all'indomani della tragedia tutti a parlare di rifugiati, poi le cose, nella discussione anche a livello europeo, vanno diversamente. Queste sono le questioni che abbiamo di fronte e che stanno a cuore a noi come Paese.

fortissima in Afghanistan, per capire cosa succede. Purtroppo i segnali sono tutti negativi, non sono positivi per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, la tutela e la difesa dei diritti delle donne, che si stanno opponendo coraggiosamente. Ricordiamo Ricordiamo quello che sta accadendo: tantissime donne stanno scendendo in piazza, sfidando con i loro corpi i talebani e noi non possiamo fare come abbiamo fatto con le donne curde, che hanno combattuto con noi contro contro i terroristi e poi sono state lasciate sole durante l'assedio. Questo è il problema. A maggior ragione oggi dobbiamo non solo attivare

unicamente se rafforziamo una capacità di vera condivisione all'interno dell'Unione europea, affinché l'Unione europea si muova in modo assolutamente unitario. La storia dirà

assolutamente più procrastinabile una capacità vera di stare in campo dell'Unione europea, e non solo in termini di difesa, questo lo vorrei rimarcare con forza. Serve innanzitutto una politica estera dell'Unione europea, la difesa viene dopo: senza la politica estera comune

rappresentano il Governo, Di Maio e Guerini, un apprezzamento per come si è comportata l'Italia, per come si è comportato il Governo italiano, sia per aver governato diligentemente e con coerenza il rimpatrio, sia per aver offerto disponibilità all'accoglienza, e voglio aggiungere infine, anche per il tentativo pressante di organizzare con rapidità un G20 straordinario sul tema oggetto anche delle nostre considerazioni. I miei apprezzamenti, signori Ministri, terminano qui. Se veniamo alla vicenda relativa all'Europa, faccio mie le considerazioni fatte, in maniera decisamente e naturalmente molto più paludata, dal Capo del Governo e dal Capo dello Stato, ma che oggi ho sentito riecheggiare anche con delle proposte interessanti da parte del Ministro della difesa. Le faccio mie insieme alle considerazioni del Ministro degli esteri. Non possiamo accontentarci di ciò che abbiamo visto. Serve molto di più. Un'Europa che non sia un soggetto geopolitico di fronte ai tornanti della storia quando la storia si avvita non è più assolutamente tollerabile. Non è più tollerabile perché la considerazione che sta a monte di questa valutazione si lega al fatto che l'America gendarme del mondo non esiste più. Ed è un errore considerare "il non esiste più" iniziato soltanto con il presidente Trump, in quanto già con la Presidenza precedente quella linea era stata marcata e irrobustita dal Presidente che ha preceduto Biden e a oggi è stata confermata. Faremmo un errore se non valutassimo che ci troviamo nel pieno di una nascente seconda guerra fredda, dove nella sfida fra Stati Uniti e Cina si sommano ambizioni di potenze regionali che rischiano di portare il multilateralismo a una condizione in cui l'Europa rischia di essere perfettamente emarginata. È già stato detto e io lo sottolineo: ogni politica di difesa in ogni tempo è sempre stata figlia di una politica estera; è la politica estera la madre, dalla quale segue una politica di difesa. il numero uno della politica estera europea, un caro amico, Josep Borrell, sostiene che deve essere costituita rapidamente una forza di pronto intervento ha ragione. Tuttavia, se non facciamo precedere la nascita di quella forza da una politica estera comune e da un orientamento che porti a una sorta di Stati Uniti d'Europa, con un'unica politica fiscale e un'unica politica estera, temo che le forze di pronto intervento

preventiva, ossia se l'Unione europea, non così come oggi la conosciamo, ma nelle dimensioni che oggi conosciamo, possa essere considerata la risposta più efficace, cioè se l'Unione europea a 27 abbia le caratteristiche per giocare una sfida che è diversa da quella giocata nell'Ottocento e nel Novecento.

Ho letto delle risposte che non stanno né in cielo, né in terra. La democrazia è sempre stata esportabile, ma non ovunque e nemmeno con la stessa velocità.

Dimentichiamo troppo spesso che la larghissima maggioranza dei Paesi del mondo ha siglato nel 1948 la Dichiarazione universale dei diritti umani. Dimentichiamo che nel settembre 2000 le Nazioni Unite hanno sottoscritto sottoscritto quasi all'unanimità una nota nella quale si diceva, testualmente, che la democrazia è un valore universale, ma non c'è un unico modello di democrazia, come è evidente. C'è un punto, però, su cui tutti siamo d'accordo: l'universalità dei diritti fondamentali non è un mito, è un diritto dei popoli. Se vengono infibulate 150 milioni di ragazzine o si impiccano gli omosessuali, la questione riguarda anche noi e l'esportabilità

che l'Italia, con questo Governo, e l'Europa possono svolgere, io mi auguro possa essere anche questa.

ancora una volta la sua gratitudine alle nostre Forze armate, ai diplomatici e a tutti coloro che, a vario titolo, hanno lavorato per la riuscita dell'operazione Aquila Omnia. Fratelli d'Italia non può tuttavia non ripetere e non stigmatizzare il ritardo registrato dal Governo, già prima

riprese abbiamo fatto affinché il presidente Draghi venisse in Aula a tenere comunicazioni con voto per indirizzo politico, perché è proprio questo che dobbiamo fare, condividere cioè un indirizzo politico su che cosa fare in Afghanistan e su come gestire gestire chi è arrivato, chi è riuscito a fuggire e deve costruire il futuro e come gestire il dramma dei profughi che, secondo noi di Fratelli d'Italia, deve essere affrontato sostenendo i Paesi confinanti con l'Afghanistan. Quando lo abbiamo detto siamo stati

perché non c'è stata chiarezza e mi dispiace anche registrare un senso di mollezza e di lentezza della politica rispetto alla velocità e alla violenza del dramma afghano. Fratelli d'Italia non intende dialogare con il regime dei fondamentalisti islamici, né intende confrontarsi con chi vuole costituire un Emirato islamico

condivisa e lo dimostra il fatto che l'Europa non è stata in grado di ragionare per tempo sulle conseguenze del terremoto geopolitico che avrebbe evidentemente provocato il ritiro dall'Afghanistan ed è assai strano che tutto ciò abbia colto molti di sorpresa, anche perché, purtroppo, non mancano precedenti negativi sulla destabilizzazione e sulla scia del caos lasciato dal ritiro

con chi non le vuole in Parlamento, con chi non le vuole medico o giudice, né le vuole far uscire da sole o viaggiare. Nessun dialogo è possibile perché, sia chiaro, non dipende da quello che faranno e da quello che diranno: sono nemici delle donne, sono nemici dei bambini, sono nemici dei diritti umani fondamentali che abbiamo insieme sottoscritto - quasi tutti i Paesi del mondo, tranne gli Stati Uniti - anche nelle convenzioni dell'ONU. Quando dunque dunque pensiamo a quanto è stato fatto, dobbiamo essere chiari. Siamo all'anno zero: questo in Afghanistan è l'anno zero che annulla tutti i successi

sapete perché? Perché è questo che i talebani odiano, il cervello delle donne e di chi non la pensa come loro.

nel ringraziare i Ministri per le loro informative, per il lavoro svolto in questo periodo, partirei dall'esercizio che è stato fatto anche da molti commentatori, forse in maniera affrettata e superficiale, definendo un fallimento gli ultimi vent'anni in Afghanistan. Penso che quando si parla di questi temi bisognerebbe approfondire, studiare, capire la complessità di quel teatro. Non desidero scomodare i tempi del *great game*, ma sia nella dimensione nazionale (il concetto stesso di Afghanistan), sia in quella religiosa dell'Islam*,* si conoscono delle faglie che sono certamente da studiare e da approfondire. Chi è stato sul posto sa che uno si sente tagico, si sente uzbeko, si sente *pashtun,* si sente *hazara*, non si sente afgano. Lo stesso Islam viene interpretato all'interno dello stesso mondo sunnita in maniera differente: i maggiori nemici sono sunniti fondamentalisti, lo scontro è tra i talebani e l'ISIS-K. Noi abbiamo operato in quel terreno e la consapevolezza della società afgana, dei propri diritti, del fatto che si possa vivere in maniera diversa, l'hanno assunta grazie a noi, grazie alla coalizione internazionale, ai militari presenti che hanno permesso alla società afgana di germogliare e di crescere, così come le stesse organizzazioni non governative hanno potuto fare il loro lavoro. Noi siamo orgogliosi di essere quel Paese che a Herat ha permesso di avere il più alto tasso di alfabetizzazione per le donne e le bambine, che per la prima volta sono potute andare a scuola, studiare e crescere nella

ha fatto a nome di tutti e di tutto il Governo il ministro Guerini quando è stato a Herat, quindi lasciamo stare le polemiche sulla Folgore e uniamoci nel ringraziamento e nel sentito applauso alle nostre Forze armate, che sono state doverosamente ringraziate e accolte Adesso ci sarà probabilmente il G20 straordinario, che non sarà facile. Penso che quello sia il luogo in cui l'Italia può giocare la sua parte, avendo la presidenza di turno. Considero corretto il viaggio che ha fatto il Ministro, operando quindi sul canale

5.000 persone, siamo orgogliosi del lavoro fatto, ma molte persone restano lì, molte persone sono rifugiate, sono nei campi, sono già *displaced people,* hanno bisogno di essere supportate e aiutate. Il G20 può essere il luogo in cui noi troviamo questi accordi, utilizzando in maniera intelligente ed equilibrata la leva degli

una recente visita negli Stati Uniti) il fatto che il rapporto nell'Alleanza atlantica è fondamentale. Ritengo che la NATO possa avere un futuro nel momento in cui avrà un pilastro europeo forte e credibile. L'autonomia strategica europea non può essere un *dossier* che apriamo a fasi alterne; è un tema che c'è, ma se lo vogliamo affrontare seriamente non può essere quello di interviste in cui annunciamo una forza di intervento rapido con 5.000 persone. Si tratta di una situazione molto più complessa, come avete detto bene nei vostri interventi. Serve un'agenda politica comune, serve capire se il nostro posizionamento è più verso il Mediterraneo, il Sahel e i Balcani o è verso la Russia. Riusciamo a contemperare le esigenze dei diversi Paesi europei e a costruire un'agenda politica comune?

non funzioneranno, perché ci vuole l'unanimità e probabilmente le cooperazioni rafforzate servono fino a un certo punto. Ma se vogliamo veramente incidere, avere una difesa europea comune, dare più forza alla NATO e giocare la nostra parte nella stabilità e nella sicurezza internazionale, serve una politica estera comune e di difesa comune. Forse lo faremo con un nucleo di protagonisti e di pionieri, come fu all'inizio quello dei Padri fondatori. Questa è una riflessione seria che va fatta, se vogliamo giocare un ruolo come Italia all'interno della Conferenza sul futuro dell'Europa e nei consessi principali. Un'ultima considerazione che riguarda un po' anche la nostra società e le società europee: tutti si sono mobilitati, giustamente, nelle piazze italiane ed europee a difesa degli afghani per la tutela dei diritti umani, dei diritti delle donne e dei bambini.

anche a morire per quei valori e per quei principi? Perché se non ci diamo questa risposta rischiamo di essere velleitari, a scendere in piazza per i diritti senza essere poi conseguenti, e dentro gli scenari internazionali conta anche l'opzione della forza, l'opzione militare. Da questo punto di vista serve una consapevolezza in più da parte dei politici che alle opinioni pubbliche dicano la verità: se vogliamo essere protagonisti in Libia, se vogliamo essere protagonisti nel Mediterraneo

Signor Presidente, non si poteva avere un epilogo peggiore di questo, dopo vent'anni di occupazione NATO, dopo vent'anni di imperialismo dei diritti umani, per dirla come Tony Blair, di retorica sulla guerra umanitaria e sull'esportazione della democrazia.

non hanno lasciato dubbi su quali erano gli interessi dell'America e non erano certo quelli di combattere una guerra altrui in casa altrui. Cosa resta? Cos'è tutta questa meraviglia, questo strapparsi le vesti? Cosa vi aspettavate? Davvero qualcuno aveva creduto che l'accordo con i talebani, sottoscritto da Trump nel febbraio 2020, ma già pensato da Obama - com'è stato detto - e poi eseguito da Biden (quattro paginette striminzite, ci dicono), avrebbe assicurato diritti e pace? Sembra che di quelle parole non ci sia traccia in quel documento: un accordo dell'amministrazione americana fatto con i talebani, plaudito dalla NATO e da tutti i Paesi che gravitano intorno all'Afghanistan e agli interessi dell'Afghanistan, senza il Governo afghano, quello voluto dagli USA, quello che è frutto dell'esportazione della democrazia. Perché? Come leggere tutto questo se non come un fallimento e una resa? Eppure, il Sottosegretario di Stato americano assicura che gli obiettivi di guerra sono stati raggiunti. Quali obiettivi? Cosa abbiamo ottenuto con migliaia di morti e una spesa di 5.400 miliardi di euro - altro che 120 milioni - che avrebbero potuto debellare la povertà più estrema del mondo? Ma soprattutto cosa lasciamo? Lasciamo un Paese sull'orlo della guerra civile, dove tutte le speranze e tutte le promesse di emancipazione contrabbandate sono state disattese e disattese e abbandonate, dove i profughi e i profughi interni sono migliaia e non da ora, dove i giovani e non solo i giovani sono ormai devastati dalla tossicodipendenza da cocaina, la cui produzione è quadruplicata in questi anni, così come il traffico di armi, e queste sono le basi dell'economia di quel Paese. Vogliamo contrastarla oggi? Arriviamo dopo vent'anni e contrastare questa economia. Come? Cosa diremo ai contadini afghani rispetto a questo? Quello a cui assistiamo non è solo il fallimento dell'intervento in Afghanistan, ma il fallimento di un mondo di idee, ed è quantomeno curioso - e varrebbe la pena farci una riflessione - che questi vent'anni coincidano con i vent'anni del G8 di Genova. Vent'anni fa, in centinaia di migliaia avevano manifestato il senno di prima, per dirlo con le parole di Andrea Segre: vent'anni fa c'era chi sentiva già con chiarezza che nello stretto *canyon* «che divideva il mondo tra pro e contro talebani, esisteva un sentiero più coraggioso che evidenziava la miopia e la follia di quella dottrina». Furono accusati di massimalismo e utopismo irresponsabile; col senno di poi, rappresentavano invece senza alcun dubbio il senno di prima. Avrebbero dovuto non fermarsi mai neanche dopo Genova, e forse dovremmo provare a ripartire tutti da lì. Ma ora, nell'emergenza, ci vogliono innanzitutto umanità e presenza. Oltre ai corridoi umanitari, che non possono essere in alcun modo riservati solo a chi ha collaborato con noi; oltre al fatto che bisogna occuparsi dell'accoglienza, per non rimandare indietro coloro che facciamo venire, come dice Laura Marmorale a Napoli, occorrerà pensare anche a come aiutare chi è intenzionato a restare lì e a resistere, così come ha chiesto a Giovanna Cardarelli del CISDA, anche lei a Napoli durante la manifestazione del 30 agosto in favore dell'Afghanistan. Ben venga il G20, signor Ministro, ma per il momento la risposta europea non è stata né unitaria, né soddisfacente. Ribadiamo anche noi la necessità di attuare pienamente la direttiva n. 55, al fine di assicurare una tutela immediata ai cittadini afghani e provare a rimediare a tutto questo. Grazie! onorevoli colleghi, signori Ministri, la crisi afghana divampata in agosto, non certo senza avvisaglie, assomma una dimensione politica e una umanitaria, ma ciò che ancora sembra sfuggire a molti sono gli effetti a medio e lungo termine della vicenda: uno spartiacque nella politica mediorientale e negli assetti internazionali. Sarebbe troppo facile recriminare sugli errori di questi anni e su quelli di questi ultimi mesi e giorni. Segnalo solo a chi anche in quest'Aula guarda le vicende estere in modo demagogico e retorico che l'esaltazione fideistica e *a priori* del modello multilateralista della nuova amministrazione Biden si si è rivelata alla prova dei fatti una propaganda ingannevole. Sebbene la presenza occidentale e USA in particolare appariva sempre più difficilmente sostenibile in Afghanistan - e per tali ragioni accordi con i talebani funzionali a regolare il disimpegno americano vennero già siglati a Doha nel febbraio 2020 sotto la presidenza Trump - non possiamo non sottolineare l'errore nel *timing* compiuto da Biden. Detto ciò, sarebbe del tutto sbagliato approfittare di questa circostanza per dare la stura a un antiamericanismo di maniera, che non appartiene alla nostra politica estera, frutto della propaganda di Pechino, che in tema di repressione di libertà e di tutela dei diritti umani delle donne non ha nulla da invidiare ai talebani, e infatti non a caso già preannuncia per Taiwan un epilogo afghano. L'America è nostro alleato strategico e un riferimento imprescindibile del mondo occidentale al quale si possono avanzare critiche, ma sul cui rapporto non ci possono essere dubbi, né tentennamenti. Inoltre, a chi, approfittando di queste vicissitudini, critica *tout court* vent'anni di presenza occidentale in Afghanistan, ricordo che, nonostante tutto, almeno la situazione del punto di vista dei diritti era migliorata: istruzione scolastica (specie femminile), tribunali laici, diritti delle minoranze, arte e cultura, che saranno ora soggetti alla scure talebana. Certo, non abbiamo risolto, forse perché irrisolvibile, il problema di creare una vera entità statuale, poiché l'Occidente è stato sì efficiente nell'intervento militare, ma si è cullato nell'illusione che il modello della democrazia liberale potesse essere imposto dall'alto,

dando vita a una sorta di gioco dell'oca, che ci ha riportato, ben che vada, alla casella di partenza. Siamo, quindi, in presenza di una sconfitta e le sconfitte contano. Nessuno può, pertanto, pensare che sarà sufficiente trattare con i talebani, subordinando il rispetto di un po' di diritti umani e di libertà alla promessa di inserire il nuovo regime, bisognoso di risorse, nel sistema del *business*. Non sarà così. sarà così. Questa idea semplicistica è magari funzionale alla costruzione di quel grande oleodotto Est-Ovest che dovrebbe passare proprio in territorio afghano. afghano. Questa impostazione minimalista difficilmente impedirà violenze, lapidazioni sommarie, l'umiliazione femminile o l'abuso di bambine, vendute in nome di falsi precetti religiosi, che rappresentano un insulto all'Islam ancor prima che ai principi fondamentali che tutelano la persona. Dobbiamo, quindi, essere consapevoli che non sarà facile imbastire una vera interlocuzione con una nascente teocrazia del narcotraffico e che nessun dialogo sarà possibile in assenza di reali e concreti segnali di apertura, che vadano al di là delle dichiarazioni di questi ultimi giorni. Nessuna interlocuzione è possibile, se impediranno alle persone che vogliono lasciare l'Afghanistan di farlo liberamente. Dobbiamo essere fermi nel pretendere il rispetto di alcune condizioni minime per il dialogo, elencate dallo stesso alto rappresentante dell'Unione europea, Josep Borrell. Diciamo chiaramente che il nostro rapporto con i talebani non sarà semplice, anche perché sarà minato da interferenze e da interessi terzi. È evidente a tutti come alcune nuove potenze mondiali, con i loro disegni egemonici, provino a mettere all'angolo l'Occidente, dimostrando il suo declino culturale, prima ancora che economico, anche al fine di accaparrarsi lo sfruttamento di uno dei più grandi giacimenti di terre rare del mondo qual è l'Afghanistan. Le dichiarazioni del portavoce dei talebani, Zabiullah Mujahid, che, mentre chiede all'Italia di riconoscere il nuovo Stato islamico afghano (decisione che, sottolineo, non può essere assunta unilateralmente dall'Italia), rivendica la *partnership* strategica di Kabul con Pechino, testimoniano la portata della posta in gioco e le difficoltà che ci attendono. La questione afghana ci impone, quindi, di aprire una seria riflessione nella comunità occidentale, specialmente all'interno di una Europa ancora una volta divisa e in ritardo sulle grandi sfide del nostro tempo. I fatti di Kabul rischiano di creare un effetto domino in tutto il Medio Oriente e di dare la stura ai tanti estremismi della regione, oltre che a rivitalizzare alcune centrali del terrore come al Qaeda a dare spazio a nuovi attori: pensiamo al rafforzamento di Qatar, Pakistan e Turchia nel mondo musulmano e al riavvicinamento di Teheran con Kabul. Sono situazioni che avranno ripercussioni importanti e che, ad esempio, possono dare alla Cina, non solo la forza di sovvertire a proprio favore gli equilibri asiatici, ma di ottenere un vantaggio e nuovi alleati nello scacchiere globale. In Siria, ad esempio, le milizie asserragliate nell'area di Idlib plaudono alla riconquista talebana dell'Afghanistan ed Hamas progetta nuovi attacchi e un *network* di alleanze. Si stagliano così all'orizzonte sfide epocali per l'Occidente e c'è molto di più da recuperare che il prestigio, l'autorità o l'urgenza di far fronte all'arrivo dei profughi. Oggi sono in ballo la nostra sicurezza e le nostre libertà. L'Europa su tutti deve fare un salto in avanti ed è qui che, come Italia, potremo giocare un ruolo, forti dell'impegno encomiabile delle nostre Forze armate nel mondo mediorientale e mediterraneo e della percezione positiva che la pregressa storia repubblicana, la tanto vituperata Prima Repubblica ancora ci regala nell'area. Ha ragione il presidente Mattarella: la retorica dell'accoglienza in Europa si scontra con la realtà dei fatti. I prossimi mesi in tal senso saranno ancora di più una cartina di tornasole, con le dichiarazioni che giungono da molte cancellerie, Berlino in testa, volte a rigettare l'idea di stabilire quote UE per l'accoglienza dei profughi. Ma di pari passo dobbiamo sapere che la minaccia di un ritorno al terrorismo jihadista impone un più stretto coordinamento fra polizie e *intelligence* nazionali nell'Unione e che la possibilità di un flusso consistente di profughi afghani in fuga dalla brutalità dei talebani richiede regole comuni e condivise per accogliere e integrare. Il tutto senza dimenticare che resta aperto il tema dei migranti economici, su cui la nostra Nazione continua a pagare un dazio pesantissimo, nonostante i piccoli progressi ottenuti nel vertice europeo dello scorso giugno dal presidente Draghi. E senza tralasciare il fatto che a breve dovremo ritrattare come Europa le condizioni dei nostri accordi con la Turchia, che regola il rubinetto dei flussi migratori dalla rotta balcanica. In sostanza, seppur declinato in diversi modi e su più *dossier*, si pone il tema di una sicurezza unica europea, che però necessita preliminarmente di una politica estera europea e quindi della definizione di quale sia l'interesse europeo. Avere una difesa integrata significa essere attori attivi sulla scena mondiale, avere capacità di proiezione e di risposta agli eventi, consci che si può raggiungere questo obiettivo solo con una riforma in senso pienamente democratico dell'Unione. Solo con più democrazia e con meno euroburocrazia, con un approccio che metta da parte assi e interessi particolari, vi saranno i presupposti per giungere all'obiettivo e quindi passare dal voto all'unanimità al voto a maggioranza.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, ringrazio innanzitutto per la calendarizzazione di questa informativa. È importante che l'Assemblea venga informata di eventi fondamentali della politica internazionale, perché le conseguenze di crisi che ci appaiono lontane e dai contorni ancora poco chiari, hanno risvolti diretti sul nostro Paese e sul nostro mondo. La storia, anche recente, ce lo ha insegnato. Per questo sviluppare un dibattito sano, che abbia a cuore tali tematiche, deve essere una nostra priorità. Come partito, sin dagli esordi dell'*escalation* degli eventi che si sono susseguiti dopo il ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan, abbiamo espresso la necessità di dover riferire al Parlamento o alle Commissioni difesa, come è successo, per discutere della crisi geopolitica che sta investendo l'area e dei riflessi geopolitici che questa avrà nel contesto internazionale, con particolare attenzione al nostro Paese. Paese. Ciò cui abbiamo assistito e cui stiamo continuando ad assistere è uno scenario drammatico, come drammatico è da intendersi il crollo del Governo afghano e delle sue istituzioni, che con grande impegno e fatica, con ingenti risorse economiche, con capacità diplomatiche e anche con la perdita di numerose vite di nostri militari, abbiamo contribuito a costruire negli ultimi venti anni. È evidente e innegabile che quanto avvenuto in Afghanistan rappresenti una sconfitta per l'intera comunità internazionale e richieda ora un'analisi e una seria riflessione sugli errori commessi dall'Occidente, *in primis* dagli Stati Uniti d'America di Biden e, a cascata, dagli altri Paesi impegnati in Afghanistan, che hanno dovuto far fronte a una ritirata che ha consentito la repentina ripresa del potere da parte dei talebani. Tali eventi hanno evidenziato i grandi limiti delle potenze occidentali, anche in termini di capacità di previsione rispetto a quanto sarebbe avvenuto all'indomani del ritiro delle truppe. Quanto è avvenuto in Afghanistan impone al nostro Paese una seria riflessione sul ruolo che l'Italia e gli altri Stati europei rivestono all'interno dell'Alleanza atlantica. un'alleanza di cui facciamo convintamente parte, ma che forse, a causa del retropensiero di una certa parte politica, abbiamo sempre vissuto in maniera esageratamente passiva. All'interno dei confini dell'Alleanza atlantica sono rappresentati anche i nostri interessi: perseguirli, insieme al nostro alleato strategico per eccellenza, gli Stati Uniti, deve essere un imperativo per la nostra politica estera del futuro. Proprio per questo è essenziale prodigarsi nel portare con forza i nostri interessi anche in questa sede multilaterale, che nella storia contemporanea ha visto l'Italia tra i primi Paesi per impegno, risorse, uomini e vite sacrificate. È necessario ripensare l'Alleanza, con la volontà condivisa e ormai palesata di giungere ad un nuovo documento strategico della NATO, nel breve periodo. Questa deve essere un'opportunità, che non possiamo lasciar correre. Il mondo sta cambiando in fretta e le grandi sedi multilaterali di cui facciamo parte, Unione europea *in primis*, hanno un'impalcatura di regole che risultano stantie ed anacronistiche. Lo stesso impegno che tutti noi - o quantomeno una buona parte di questa Assemblea - abbiamo palesato nella volontà di riscrivere le vecchie regole economiche dell'Unione europea, superate dalla storia, dobbiamo palesarlo anche nella volontà di giungere ad un rinnovamento del concetto strategico dell'Alleanza atlantica. In questa riscrittura di regole e linee guida è fondamentale avere il coraggio di impegnarsi. L'Europa finora non è stata in grado di gestire la crisi afghana e deve ora riguadagnare una nuova credibilità nella gestione della situazione. L'Italia ha ora l'opportunità di rivestire un ruolo centrale, a partire dalla prossima riunione del G20, presieduto dal nostro presidente del Consiglio, Mario Draghi, a cui chiediamo di voler allargare la partecipazione anche a quei Paesi non invitati che possano contribuire alla serenità dell'area. Non possiamo consentire che la Cina investa, come già sembrerebbe abbia iniziato a fare, nel Paese centro-asiatico, nella sua ricostruzione e nel riconoscendo magari il Governo talebano e il neocostituito emirato islamico, sancendo di fatto il loro controllo dell'area. Non può essere di certo una soluzione quella prospettata da alcuni esponenti politici, per cui può essere preso in considerazione un riconoscimento di tale Governo da parte del nostro Paese o l'avvio di un dialogo con i talebani, illudendosi che essi possano rivelarsi diversi da ciò che in realtà sono, dimenticando le esecuzioni a cui ci hanno a cui ci hanno abituato, i nostri connazionali morti per combatterli, le condizioni medievali in cui vorrebbero far tornare a vivere il Paese e la loro considerazione delle donne. Oltre alla questione geopolitica e al ruolo che intende svolgere l'Italia nel contesto internazionale e a quelle che saranno le opportune riflessioni anche sulle altre missioni in cui siamo coinvolti, evitando l'eventualità che possa verificarsi quanto avvenuto in Afghanistan, ci piacerebbe sapere come intenda muoversi il Paese con riferimento ai rimpatri e agli ingressi in Italia. Riteniamo che si debbano assolutamente mettere in sicurezza coloro che negli anni hanno collaborato per rendere l'Afghanistan un Paese democratico e allo stesso tempo auspichiamo che la comunità internazionale intervenga rapidamente, per evitare che la fuga dai talebani si trasformi in un esodo incontrollato, che avrebbe

ora sono 2,5 milioni, stando alle ultime stime, coloro che intendono abbandonare il Paese. Senza una pianificazione seria e condivisa tra tutti gli Stati, rischiamo che le fughe si trasformino in un esodo disordinato, con enorme pregiudizio per chi fugge e per i Paesi di destinazione. Bisogna altresì scongiurare il rischio di infiltrazione terroristica attraverso l'immigrazione illegale e su questo i Servizi e le *intelligence* dovranno mostrare un'attenzione e una capacità ben superiori rispetto a quelle messe in atto

morte, droga e malori si sono susseguiti per oltre sei giorni. In uno dei tanti discorsi alla Nazione fatti durante i tragici Biden ha usato un termine significativo con riferimento alle future traiettorie del terrorismo internazionale. Ha detto letteralmente che il terrorismo si è diffuso come una metastasi nel mondo. È una visione corretta: la frammentazione e la fluidità dei grandi *brand* del terrorismo dall'ISIS ad al Qaeda è una forma di realtà conclamata. È al contempo un pericolo. I confini del contrasto al terrorismo sfumano, il pericolo cambia e devono cambiare le nostre capacità di risposta. Nel concludere, signor Presidente, ricordo che la lotta al terrorismo, iniziata nel 2001 in Afghanistan, ha messo a durissima prova la tenuta di al Qaeda, che ha sofferto l'eliminazione dei suoi principali esponenti e si è indebolita enormemente. Adesso al centro dell'Asia ritroviamo un Paese allo sbando, con al potere quegli stessi guerriglieri che diedero casa, ospitalità e risorse ad al Qaeda permettendole di infiammare il mondo. Serve grande attenzione e occorre ribadire che la priorità della classe politica italiana ed europea nei prossimi anni è quella di mettere in sicurezza il nostro Paese e il nostro continente. La storia ci ha insegnato cosa vuol dire sottovalutare i problemi; non cadiamo nello stesso errore.

Ministri, colleghi, anzitutto voglio porgere, a nome di tutto il Gruppo MoVimento 5 Stelle del Senato, un ringraziamento veramente sentito e non di circostanza ai qui presenti ministri Di Maio e Guerini per il grande lavoro che hanno svolto per portare in salvo nel nostro Paese non solo i nostri concittadini, ma anche 5.000 afghani. Grazie! Nessun altro Paese europeo si è prodigato così tanto a favore dei nostri amici afghani, e a questo proposito un particolare encomio va rivolto al diplomatico italiano Tommaso Claudi, rimasto fino alla fine a Kabul per portare in salvo quante più persone possibili. Farnesina e Difesa, con il prezioso contributo della nostra *intelligence*, hanno realizzato il massimo risultato possibile, trovandosi a operare nella peggiore delle situazioni, quella pesante eredità che anche il presidente Biden si è trovato a dover gestire, causata dalle scelte sbagliate delle passate amministrazioni statunitensi che, invece di porre fine a questa guerra dieci anni fa, quando fu eliminato Bin Laden, decisero di rimanere a oltranza per poi lasciare il Paese ai talebani, senza concordare con loro un ordinato e ben gestito passaggio di consegne del potere. Rimanere ha significato prolungare inutilmente una guerra che ha inferto sofferenze incalcolabili al popolo afghano e ai tanti militari occidentali che hanno perso la vita. Un ricordo sentito in particolare va ai nostri 54 caduti e 700 feriti. *(Applausi)*. il MoVimento 5 Stelle chiedeva la fine della guerra in Afghanistan e il ritiro delle nostre truppe da quel Paese. È stato il nostro primo atto parlamentare, la prima mozione che presentammo appena entrati in Parlamento. Dicevamo allora - e abbiamo continuato a dirlo in tutti questi anni - che quella era una guerra inutile perché non c'è mai stato un reale motivo per dichiarare guerra ai talebani afghani, i quali non solo non avevano responsabilità negli attentati dell'11 settembre responsabilità da ricercare altrove a partire dall'Arabia Saudita - ma erano anche disposti a consegnare Bin Laden, offerta che fu rifiutata dall'allora presidente George Bush, vero responsabile di questa impresa bellica insieme a Tony Blair e ai loro sodali europei, tra cui spiccava l'allora *premier* italiano Silvio Berlusconi. Dicevamo allora che quella guerra, come ha ricordato nel suo ultimo articolo il compianto Gino Strada, non è mai stata una missione di pace, ma una guerra lanciata dagli Stati Uniti senza nessuna autorizzazione da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU e quindi al di fuori della cornice del diritto internazionale e del diritto universale dei popoli all'autodeterminazione. La nostra partecipazione a questa guerra è stata infatti una palese violazione dell'articolo 11 della nostra Costituzione e di questo se ne dovrebbe assumere la responsabilità chi governava al tempo il nostro Paese. Dicevamo allora che esportare la democrazia usando la forza militare è una contraddizione di termini e infatti si è rivelato un fallimento totale. Dicevamo che questa guerra stava portando solo ulteriore distruzione, morte e povertà a una popolazione già devastata da decenni di conflitti. Affermavamo anche che invece di contrastare la produzione dell'oppio durante l'occupazione, l'Afghanistan è diventato un narco-Stato che ha inondato il mondo di eroina dicevamo allora che i trilioni di dollari spesi per distruggere l'Afghanistan a vantaggio del complesso militare-industriale potevano essere spesi decisamente meglio sia lì per la ricostruzione e lo sviluppo di quel Paese, sia qui da noi per il benessere dei nostri concittadini. Già otto anni fa, infatti, era chiaro che la guerra era persa, perché i talebani già allora controllavano di fatto la maggior parte del territorio afghano. Purtroppo per anni siamo stati inascoltati, anzi sbeffeggiati e derisi come poveri ingenui e ignoranti. Oggi, dopo che i fatti hanno smentito vent'anni di propaganda dandoci ragione, le nostre posizioni sono condivise da tutti, lo abbiamo sentito anche oggi. Mi domando e vi domando: coloro che ironizzavano sulle nostre posizioni - penso a politici, intellettuali, giornalisti - avranno l'umiltà di rendere onore alla lucidità che il MoVimento 5 Stelle ha sempre avuto su questa triste vicenda? Purtroppo temo di no. Lo dimostrano gli ignobili attacchi rivolti a Giuseppe Conte, solo per aver detto la semplice verità, e cioè che è importante tentare di instaurare un dialogo con i talebani. Attenzione, questo non equivale a riconoscerli o legittimarli, ma chi ha dimestichezza almeno con l'alfabeto delle relazioni internazionali sa che è una strada che va tentata. Giuseppe Conte è stato addirittura accusato di essere l'avvocato dei talebani, allora la stessa accusa andrebbe mossa anche all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell, all'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati Filippo Grandi, alla cancelliera tedesca Angela Merkel e a tanti altri. Il dialogo con i talebani, avviato dagli stessi statunitensi, è l'unico strumento per pressarli al fine di ottenere da loro quello che ci interessa: oggi corridoi umanitari, domani il rispetto dei diritti umani, in particolare di quelli delle donne. Potrà essere una realtà di fatto a noi sgradita, ma sono i talebani ad aver vinto la guerra e sono loro che controllano il Paese, quindi è con loro che dobbiamo tentare di instaurare un dialogo se veramente ci interessa influire positivamente sul destino del popolo afghano. Coloro che oggi dicono «mai dialogo con i talebani» sono gli stessi che fino a ieri volevano continuare all'infinito questa guerra, ma isolando quel regime sarà solo peggio, non solo per gli afghani, ma anche per noi. Se l'Occidente e l'Europa si oppongono ad un dialogo, il regime si radicalizzerà pericolosamente, finanziandosi con la *jihad* antioccidentale e con il narcotraffico, o si rivolgerà ad altri poco affidabili attori internazionali che non aspettano altro. Concludo dicendo che l'esperienza dovrebbe insegnare a tutti i presunti maestri di geopolitica che invece di attaccarci forse è meglio dare ascolto a quello che sostiene il MoVimento 5 Stelle, rendendo l'Italia e l'Unione europea protagonisti di una vera missione di pace, di una forte iniziativa diplomatica volta ad intavolare una trattativa condizionata con chi governa oggi l'Afghanistan. Aiuti in cambio di rispetto dei diritti umani, al solo scopo di alleviare la situazione della popolazione di quel Paese. Questa è l'unica via per rimediare a vent'anni di errori, lo dobbiamo al popolo afghano che non può essere abbandonato e ai tanti ragazzi italiani ed europei che per l'Afghanistan hanno sacrificato la loro vita. Esprimo grande apprezzamento per l'approccio pragmatico e le coraggiose iniziative diplomatiche illustrate poco fa dal ministro Di Maio, dal piano di azione nazionale al sostegno del popolo afghano, alla proposta di un G20 dedicato all'Afghanistan, su cui avrà il nostro massimo sostegno.

una nuova finestra"). La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito il calendario dei lavori fino al 16 settembre. Il prosieguo della settimana corrente è riservato ai lavori delle Commissioni. Il calendario della prossima settimana prevede, a partire da martedì 14 settembre, alle ore 16,30, la discussione del decreto-legge n. 105 sull'emergenza Covid-19, in corso di esame alla Camera dei deputati, nonché i disegni di legge delega sulla riforma del processo penale, approvato dalla Camera dei deputati, e del processo civile, ove conclusi dalla Commissione. La Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi martedì 14 settembre, alle ore 15. La seduta verrà ora sospesa fino alle ore 16,30 e riprenderà con la commemorazione della figura del compianto senatore Saviane. **Calendario

Senatori, desidero rivolgere un commosso pensiero al senatore Paolo Saviane, politico concreto, competente e appassionato. Paolo Saviane è stato un autentico protagonista della vita istituzionale del Bellunese e delle sue montagne, territori che conosceva bene e che in lui avevano trovato un fedele interprete e un importante punto di riferimento per la difesa delle loro peculiarità e delle loro istanze. Una sensibilità spontanea la sua, arricchita anche da tanti anni di esperienza come imprenditore nel settore dei legnami. Un'attenzione instancabile ai tanti problemi di ogni giorno delle comunità montane, che ha contraddistinto ogni fase del suo percorso al servizio dei cittadini. Un percorso che Paolo Saviane aveva iniziato nel 2012 con l'elezione al Consiglio comunale di Puos d'Alpago, città dov'era cresciuto, e che dopo tanti anni come segretario della Lega Nord nella provincia di Belluno stava proseguendo con impegno e dedizione da senatore in questa legislatura. Ho ancora chiaro il ricordo di uno dei suoi ultimi interventi in quest'Aula, in occasione della discussione generale sul decreto-legge in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri: un'esortazione sincera e sentita a far sì che l'istituzione di un Ministero per la transizione ecologica potesse davvero tradursi in nuove e migliori politiche pubbliche per tutelare l'ambiente, valorizzarne le ricchezze, renderlo una opportunità per le generazioni di oggi e quelle future. La malattia, con cui combatteva con tenacia da tempo, non ne aveva mai scalfito il sorriso, la voglia di fare, la disponibilità a a rimboccarsi le maniche e quel non comune senso di responsabilità nei confronti dei cittadini, che era da sempre una delle sue più forti virtù. La notizia della sua improvvisa scomparsa è stata motivo di grande dolore per tutti. Con Paolo Saviane perdiamo un collega leale, una bella persona, sempre disponibile al confronto sincero, aperto e costruttivo, nel rispetto delle posizioni e del pensiero di tutti. Rinnovo pertanto il mio cordoglio e la mia personale vicinanza al dolore dei familiari, dei parenti e degli amici del senatore Paolo Saviane.

Si potrebbe parlare molto di Paolo Saviane, forse proprio perché lui parlava molto poco. Era un uomo nato e vissuto in montagna, nella sua montagna, quella di Alpago, e di quel territorio era figlio, tanto che ne aveva assunto la concretezza, la sincerità e la semplicità. Non è stato solo un senatore, un politico, un dirigente di partito, ma anche un bravo e serio imprenditore. Nacque in una famiglia numerosa e seguì subito le orme della stessa, lavorando nella segheria del padre, che contribuì poi a sviluppare con i suoi fratelli. Spesso nei viaggi in treno mi ricordava i primi tempi in cui i vecchi andavano a tagliare le piante in bosco, mi spiegava il nome degli utensili e le modalità che si usavano. Del mondo del legname Paolo parlava con passione, spesso con apprensione; ne conosceva i sistemi e ne aveva vissuto direttamente anche i periodi più difficili. Pensava anche oltre in merito al legno e rifletteva sul futuro di un settore che ha patito una grande crisi. Paolo contribuì anche a fondare un consorzio di impresa e il relativo marchio, Legno Veneto, e di quel legno veneto in altro modo ne parlò spesso dopo il terribile tornado Vaia che lasciò molto di quel legname per terra. Del Veneto era orgoglioso e al suo territorio era legato da un sentimento indissolubile. Fu consigliere comunale, consigliere della comunità montana e fin da subito interpretò il suo ruolo non come un fine, ma come un mezzo per promuovere la sua terra e per dare ad essa un futuro. Fu anche per certi versi precursore di progetti che solo anni dopo divennero argomento di discussione. Nel programma delle elezioni comunali del 1995 parlò addirittura di un progetto di fusione di Comuni al fine di unire le forze di quelle piccole realtà montane spesso sofferenti. La passione, la innata prudenza e l'equilibrio lo hanno poi portato a rivestire ruoli prima all'interno della Lega, come segretario provinciale di Belluno, e poi come senatore.

La montagna non l'ha mai dimenticata e tutta la sua azione parlamentare la incentrò sulla questione degli impianti sciistici, per le iniziative *post* tornado Vaia o per il riconoscimento della ZES nelle zone montane. Lo abbiamo conosciuto così: un mediatore di natura, un uomo rasserenante e disponibile, un uomo così per bene che chiedeva scusa anche quando aveva ragione. La sua bontà e la sua gentilezza non gli hanno mai fatto venire per nulla meno la determinazione e la caparbietà che dimostrava nel lavoro. Era veramente di poche parole, ma anche di tanti fatti. Anche per queste ragioni, io stessa, quando ero Ministro degli affari regionali e delle autonomie, nel 2018 gli ho conferito il mandato di delegato nel Comitato dei fondi dei Comuni di confine: un incarico che ha portato avanti con lealtà ed equilibrio, con dialogo continuo con i sindaci, in un confronto con e tra gli enti e i territori che, mai più di oggi, è essenziale nell'azione politica. Era veramente orgoglioso di quel mandato, ma solo perché gli permetteva di lavorare e di dare risultati concreti a quella montagna che era la sua radice, il suo principio, ma anche il suo fine. Paolo, ti ha tradito il cuore, il cuore che era la tua forza. l'affetto di tutti voi, colleghi senatori, mi permetto di ringraziarvi, a nome nostro e della famiglia, per tutti i messaggi che ci avete mandato. La ricchezza, l'energia e la volontà di un uomo, però, sopravvivono anche a lui stesso. Noi colleghi lo porteremo sempre con noi. Sei e resterai per sempre un uomo leale, un amico sincero, un servitore delle idee e non degli uomini e un bravo leghista. Ciao, fratello.

Due brevi parole anche da parte mia, a nome del Gruppo per le Autonomie, per associarmi al dolore per la scomparsa del caro amico, senatore Paolo Saviane, e porgere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e al Gruppo della Lega. Molto brevemente, anche lui, come noi del Gruppo per le Autonomie, era un uomo di montagna, un fiero un fiero rappresentante delle Alpi bellunesi. Spesso ci trovavamo a discutere delle problematiche e delle necessità dei nostri territori. Lui faceva parte, in modo molto competente,

era una persona calma, educata e soprattutto molto competente. Il suo modo di essere era quello di un uomo riservato e parco di parole, ma, quando parlava, sempre saggio, appassionato, schietto, con un amore sviscerato per la sua terra e sempre con l'obiettivo del bene della sua gente. Se n'è andato in punta di piedi, dopo una lunga malattia che ha sorpreso, credo, non solo me, ma quasi tutti in quest'Aula. Se n'è andato con la riservatezza dei montanari. Prima, quando c'è stato il ricordo del Presidente, non ho partecipato all'applauso, come si fa da noi, gente di montagna, quando salutiamo la solennità della morte con il silenzio e la riflessione. Ciao Paolo, adesso riposa in pace. Signor Presidente, è difficile intervenire dopo le parole della ministra Stefani. Ricordare il collega Paolo Saviane è davvero difficile in questo momento, perché è stato per tutti noi una persona veramente disponibile, con la quale si diventava subito amici, anche se era di poche parole. È scomparso purtroppo troppo presto, a causa di una lunga malattia. Come è stato ricordato, faceva parte della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato e si era sempre dimostrato vicino e portavoce delle esigenze delle realtà montane, talvolta dimenticate, del Veneto e non solo,

Dispiace moltissimo, non solo perché avrebbe avuto tutta la vita davanti per sviluppare i progetti cui lavorava da anni, ma anche per la grande stima che noi tutti nutrivamo e che continuiamo a nutrire per lui. Abbiamo perso davvero un collega gentile, disponibile, un punto di riferimento, in primo luogo per la realtà dalla quale proveniva, quella bellunese. Con Paolo Saviane se ne va un politico capace, vicino al territorio, che ha sempre nutrito una grande passione per la politica e per la sua terra, che ha cercato di valorizzare, non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale, da senatore. Si è sempre messo a disposizione delle amministrazioni locali e del territorio, con quello spirito di servizio che ha continuato a dimostrare anche quando è arrivato in Senato; sempre disponibile al dialogo, a confrontarsi. Ricordo che qualche volta ci siamo ritrovati in treno, insieme alla ministra Stefani, a dialogare proprio di quegli argomenti che erano a lui più cari, a partire proprio dalla Regione Veneto. Veneto. Voglio ricordarlo anch'io così, come una persona per bene, che ha lasciato sicuramente un'impronta importante. Rivolgo le più sentite condoglianze mie del Gruppo Italia Viva-PSI alla famiglia, a tutti coloro che gli sono stati vicino e ai colleghi e alle colleghe della Lega.

Devo dire che Paolo, insieme ad altri colleghi, ha mostrato molta attenzione, ma soprattutto rispetto per questa proposta della Regione Sicilia, rispetto che non ho notato assolutamente nella

figurano nelle reti televisive e a livello comunicativo; ebbene, egli era, come altri hanno già affermato, una persona concreta, di fatto, discreta. Penso che questo, a livello politico, debba servire a tutti come esempio. L'esempio deve essere quello di un sistema valoriale di fondo, che vada al di là delle divisioni partitiche e che veda come obiettivo il bene comune e la *res publica*,

Quando un politico giunge invece ad attaccare e ad aggredire verbalmente, anche sul piano personale, un altro collega, significa che è privo di contenuti. era invece sempre sui contenuti: era un confronto autentico. Concludo dicendovi che il giorno che è arrivata la notizia della morte di Paolo Saviane mi trovavo a dover gestire una giornata lieta, un compleanno, e

Signor Presidente, nel suo intervento e nelle parole della ministra Stefani è stata riassunta l'esperienza di vita e l'impegno politico del collega Paolo Saviane, imprenditore del legno e quindi persona estremamente concreta e attenta alle esigenze di chi lavora. Presidente del Consorzio Legno veneto, consigliere dell'Unione montana, consigliere comunale di Puos d'Alpago, segretario della Lega. Come è stato ben ricordato, che tutte queste esperienze traducano le due cifre distintive della sua esistenza e della sua vita: territorio e politica. Sono due parole, un binomio, che non dovrebbe mai essere scisso per chi, come noi, si occupa della cosa pubblica. lo ha fatto con uno stile, come tutti hanno ricordato, davvero particolare. Tutti hanno riconosciuto la sua educazione e il suo approccio sempre corretto, gentile e disponibile al confronto.

Il Presidente ha ricordato il suo ultimo intervento, qui in Aula, in cui si era occupato di una questione specifica, ma potrei ricordare quando in Commissione finanze e tesoro si è discusso dei ritocchi alla legge sulle banche di credito cooperativo, banche del territorio, oppure i provvedimenti in Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, che hanno avuto a che fare con i temi della montagna o del legname. che ha davvero dedicato tutta la sua esistenza a ciò che gli era più caro: la propria terra, il proprio territorio e la propria gente. Credo che sia un esempio bello e, come purtroppo spesso accade quando qualche collega ci lascia, siamo tutti chiamati a riflettere su questi aspetti e su questi fatti: se quando siamo operativi, in vita, le persone si accorgano e apprezzino veramente ciò che facciamo e lo stile che usiamo. Riconoscerlo quando non ci siamo più è certamente una cosa bella e importante, però vorrei che questo aspetto fosse riconosciuto anche mentre ciascuno di noi opera. Paolo Saviane - tutti lo abbiamo detto - è riuscito a far brillare queste sue doti e queste sue capacità. A nome dunque del Gruppo Partito Democratico rinnovo quindi, anche da parte nostra, la vicinanza ai familiari, al Gruppo Lega e a tutte le persone che gli hanno voluto bene.

anche a nome di LeU-Ecosolidali e di tutti i membri del Gruppo Misto voglio esprimere il più profondo cordoglio e sincera vicinanza ai familiari, agli amici e ai colleghi della Lega

qualità umane, già più volte ricordate. Questo è segnale chiaro dell'universalità del giudizio che ciascuno di noi ha avuto di Paolo, che ha tutt'ora e che conserverà nel ricordo, di disponibilità, di correttezza, di educazione, di confronto e di competenza. Paolo probabilmente rappresenta uno dei modelli ideali di parlamentare, di chi rappresenta la nazione e allo stesso tempo in maniera appassionata e competente difendeva la sua terra, il suo Veneto, il suo Bellunese, la sua montagna, che ha fatto quasi amare anche a chi, come me, uomo del Sud, ha poca confidenza con quei territori. Di Paolo rimarrà in tutti noi un ricordo indelebile e ci ricorderemo di lui tutte le volte in cui la passione politica, lo scontro e il confronto dialettico rischieranno di farci perdere un po' il controllo, di andare sopra le righe. Paolo era di una pacatezza pari alla sua disponibilità e intelligenza. Paolo veramente sarà con noi e lo ricorderemo tutti come collega competente e appassionato, soprattutto dal punto di vista umano per chi ha avuto modo di conoscerlo nel breve tempo di frequentazione di questa assise. Riposa in pace. Rinnovo le condoglianze e la vicinanza a tutti coloro che Paolo ha amato e dal quale hanno ricevuto amore. Presidente, colleghi, ho chiesto alla mia Presidente di Gruppo di parlare a nome di Forza Italia perché la sua dipartita improvvisa mi ha colpito profondamente. Non conosco tutta la sua vita che lei, Presidente, ha riassunto poco fa. Il fatto di non conoscere le nostre vite e le nostre esperienze è un limite di tutti noi tra di noi perché, se conoscessimo le nostre vite, forse sarebbero diversi i rapporti e le storie. Tre anni di amicizia sono importanti. Ci raccontavamo a spicchi i fatti, le esperienze e le aspettative di essere qui in Parlamento come senatori. Era un uomo vero e parlo di uomo nell'accezione onnicomprensiva di uomo e donna. Era educato e discreto; di poche parole, ma quelle poche erano sagge ed efficaci, riassuntive ed esplicative della società, dei suoi bisogni, delle sue sensazioni e delle speranze. Sono stato - credo - tra gli ultimi a parlargli prima che fosse impossibilitato a presenziare perché non stava bene e doveva fare delle visite. Traspariva timore dai suoi occhi, ma anche una speranza. Disse: ci troveremo ancora per momenti di festa.

Si dice sempre che se ne vanno i migliori. In questo caso è proprio vero. Questa Assemblea perde qualcosa di impalpabile, di commovente e di costruttivo. perciò, un ricordo forte, una speranza, una certezza, un impegno verso la sua famiglia, verso il collegio, tutte le persone che rappresentava una volta che si è eletti e verso il Gruppo Lega. Per chi vuole rivolgiamo anche una preghiera.

Si è approcciato subito con timidezza, ma con voglia di fare e di interagire per il suo territorio, per la politica. Era un uomo mite; ogni tanto ti guardava, ti sorrideva e gli sorrideva tutto il volto. Ti accoglieva e si faceva accogliere in quest'Aula e nelle Commissioni dove - come spesso si è detto - si arriva allo scontro. Ebbene, lui ci ha dato un esempio di come la politica si può fare ascoltando, confrontandosi lavorando assieme. Abbiamo portato avanti il disegno di legge su Chioggia tutti insieme, e lui è stato parte attiva con tutti gli altri

Quando ho saputo la notizia, ho cercato di parlare con i colleghi della Lega perché mi sembrava inverosimile

Cerchiamo di non dimenticarlo mai, perché ci ha dato un grande esempio di politica e di umanità. *(Applausi)*. Ringrazio a tutti per questo momento di grande partecipazione e di commozione per il nostro collega scomparso.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

Signor Presidente, lo scorso 2 settembre si è celebrato il centenario della morte di Napoleone Colajanni, giovanissimo garibaldino appena quindicenne, docente universitario, sociologo e saggista ennese, la cui attività politica, iniziata nel 1872, lo vide consigliere comunale nella sua Castrogiovanni (l'attuale Enna), consigliere provinciale fino al 1890, quando divenne deputato alla Camera del Regno, rieletto successivamente per dieci legislature, fino alla sua morte. Guida dei repubblicani in Parlamento, fu vicino al movimento dei Fasci dei lavoratori siciliani, sposando la causa sociale del proletariato urbano, di braccianti agricoli, minatori e operai, mediando con il Governo Crispi per evitarne la repressione. Promosse importanti iniziative parlamentari come l'inchiesta sull'Eritrea, ma Napoleone Colajanni sarà ricordato come colui che fece scoppiare lo scandalo della Banca Romana, denunciando in Parlamento il perverso intreccio del malaffare tra politici e banchieri. Grazie alla sua concezione morale ed etica della politica, l'Italia intera, il 20 dicembre 1892, poté scoprire gli ammanchi milionari di una banca pronta a foraggiare imprenditori, politici e perfino le più alte cariche dello Stato. La sua denuncia portò, un mese dopo, all'arresto del governatore della Banca Romana e successivamente alle dimissioni di Giolitti da presidente del Consiglio. Come medico e criminologo avversò le teorie lombrosiane, affermando che il delinquere traeva origine da fattori ambientali e socio-economici e su questi ultimi centrò i propri studi. Nel 1898 pubblicò un opuscolo dal titolo «Per la razza maledetta», con la quale intese confutare la concezione razzista di Cesare Lombroso. Si intestò la causa dei lavoratori del latifondo siciliano e dei carusi, i giovani operai delle miniere di zolfo, proponendo la diffusione della cultura e la presa di coscienza politica delle masse come strumento per il riscatto morale e civile dell'Isola e del meridione. Straordinaria figura, non sufficientemente studiata, Napoleone Colajanni concluse il suo saggio sulla mafia con queste parole: «Il regno della mafia in Sicilia non cesserà se non il giorno in cui con una vera *instauratio ab imis* i siciliani acquisteranno la libertà vera, il diritto e i mezzi di punire i prepotenti, di mettere alla gogna i ladri e di assicurare a tutti la giustizia giusta». Presidente, alla ripresa dei lavori dell'Assemblea sento il dovere morale e civico di ricordare un mio concittadino tanto illuminato e acuto, un uomo delle istituzioni che ha lottato in favore delle masse e contro i mali che affliggevano il Paese. Ancora oggi quelle piaghe denunciate a gran voce da Colajanni creano le distorsioni politiche e sociali nelle quali prosperano illegalità e malaffare, spesso con il silenzio dello Stato, in uno scenario - diciamolo sinceramente - non diverso dal passato.

Vorrei ora soffermarmi su una crisi aziendale per esprimere solidarietà e sostegno alle preoccupazioni espresse dai sindacati e dai sindaci del Sangro, dell'Aventino e della zona frentana, per affrontare la questione della Sevel Stellantis. preoccupazioni sono state anche formalizzate ai ministri Giorgetti e Orlando da parte delle organizzazioni sindacali che sollecitano Stellantis ad alzare il velo sulle sulle proprie intenzioni prima che vengano messe nero su bianco nel nuovo *business plan*, anche per arginare gli impatti lavorativi provocati dalla carenza di approvvigionamento dei semiconduttori prodotti in Malesia. Credo non sia solo questione di *microchip*. Ad inizio 2022 sarà presentato il primo piano industriale di Stellantis ed è legittimo, stante l'attuale situazione, ipotizzare un intervento sulla sulla forza lavoro, sulle fabbriche, per riuscire a centrare i *target* della fusione, mentre i siti produttivi dei singoli Paesi dell'impero FCA e PSA si fanno concorrenza portando ognuno avanti le proprie rivendicazioni. Sappiamo anche che l'*automotive* fa i conti con la transizione ecologica del mercato delle quattro ruote, la riconversione di interi comparti dell'indotto e una fusione in corso appunto tra FCA e PSA; operazione che già al momento del varo presentava alcune criticità, sovrapposizioni, sovraccapacità produttiva, un ammontare dei costi complessivi superiori a quelli delle fabbriche spagnole e francesi. In Val di Sangro, dove si assemblea il Ducato come veicolo di punta, il mezzo più venduto in Europa, sito dove si lavorava anche per la concorrenza con Peugeot e Citroen, la produzione di 300.000 furgoni rischia di venire condivisa e calibrata al di sotto delle richieste di mercato; un ridimensionamento questo che potrebbe impattare sull'occupazione diretta e sull'indotto industriale della componentistica. La situazione produttiva della Sevel è caratterizzata da grande incertezza per tutti i lavoratori a partire dagli interinali e *staff leasing*. Non è mai successo nella storia di FCA e FIAT che il livello occupazionale del personale interno fosse così basso rispetto al numero dei lavoratori somministrati, che invece sono in numero elevatissimo e per un periodo così lungo. Nei mesi scorsi l'azienda è stata sollecitata ad assumerli; si ipotizza una ad assumerli; si ipotizza una perdita di circa 700 posti di lavoro. Sappiamo anche che lo stabilimento in Val di Sangro sta subendo la concorrenza del sito polacco di Gliwice dove si produceva l'Opel Astra,

denunciano i sindacati - intere fiancate del furgone da assemblare oltre confine e alcune aziende dell'indotto abruzzese stanno già producendo per lo stabilimento polacco, aprendo *in loco* nuove fabbriche anche per sfruttare la decisione di Varsavia di estendere nell'area gli incentivi fiscali della ZES, l'elevata infrastrutturazione di una zona strategica per servire tutto il mercato europeo. La ZES polacca prevede tantissime agevolazioni e anche deroghe

Questa interrogazione riguarda la riapertura della discarica di Roncigliano ad Albano laziale, già individuata dal ministro Cingolani come una soluzione vari mesi fa e poi riaperta tramite una ordinanza contingibile e urgente da parte della sindaca Raggi prima e poi tramite un'ordinanza del presidente Zingaretti. Ebbene, quella discarica era chiusa da tempo perché nel 2016 aveva preso fuoco l'impianto TMB ed erano stati conclamati i danni ambientali che questo aveva causato. Era chiusa da tempo perché nella zona sotto la discarica l'incidenza di tumori è molto più alta rispetto ad altre zone e rispetto alla media nazionale, sono stati rilevati metalli pesanti e inquinanti al di sopra dei limiti delle acque ad uso umano, gli abitanti della zona sottostante non hanno neanche l'acqua corrente, ma hanno solo i pozzi. È una zona agricola di grande pregio. Sulla discarica pendeva un'interdittiva antimafia che avrebbe consigliato di non riaprirla così tal quale, ma prima di verificare se le ragioni che avevano portato all'interdittiva fossero decadute, esiste un'autorizzazione di impatto ambientale scaduta dal 2009, rinnovata in maniera surrettizia e inopportuna da parte di una dirigente della Regione Lazio, che è stata a lungo ai domiciliari proprio per le accuse di concussione e corruzione riguardo ad un'altra discarica. I dati ARPA sui rifiuti sversati dimostrano che il 50 per cento dei rifiuti arrivati a quella discarica non sono a norma. I cittadini sono in presidio permanente da agosto e nessuno è andato ad esprimere loro solidarietà e nessuno risponde riguardo a queste illiceità.

anche in ottemperanza dell'impegno che tutti abbiamo profuso nel PNRR per la transizione ecologica, che perlomeno il Ministro venisse a rispondere ad un'interrogazione sul suo operato e sull'operato degli enti locali riguardo a questa discarica. La ringrazio, Presidente, di avermi concesso di parlare nonostante non fossi iscritta. **Atti e